apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Nella seduta di oggi saranno discussi i disegni di legge concernenti l'istituzione del Museo della Shoah in Roma (dalla sede redigente) e le disposizioni sanzionatorie per il deturpamento dei beni culturali e paesaggistici. A partire dalla seduta di domani saranno posti all'ordine del giorno i seguenti provvedimenti dalla sede redigente: diffusione telematica di contenuti tutelati dal diritto d'autore, approvato dalla Camera dei deputati; Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza; agricoltore custode dell'ambiente e del territorio; istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria; ripristino della festività nazionale del 4 novembre. Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del disegno di legge sul divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Gli emendamenti dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi parlamentari del testo approvato dalle Commissioni riunite. Giovedì 13 luglio, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri del lavoro, della salute e per gli affari regionali. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché del decreto-legge sugli enti territoriali, l'attuazione del PNRR e il settore energetico, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Giovedì 20 luglio, alle ore 15, si svolgerà il *question time*.

mentre noi eravamo in Conferenza dei Capigruppo, il ministro Fitto ha comunicato all'esterno, al Paese, alla stampa,

senza comunicare quali, ma di fatto ha ammesso quello che le opposizioni più volte hanno sottolineato in quest'Aula, quello che il Partito Democratico aveva denunciato, e cioè che la quarta rata non è più certa. Sicuramente non è certa nel 2023. Questo non solo ci indigna, ma ci preoccupa, perché è una navigazione a vista

Non è possibile, signor Presidente, che siamo nella condizione di partenza e oggi prendiamo atto degli esiti della riunione della cabina di regia, riunita d'urgenza probabilmente perché oggi la stampa era unanimemente critica sulla condizione del Governo italiano rispetto alla gestione del PNRR. Il risultato della cabina di regia è che il Paese prende atto che la quarta rata non c'è più o, se c'è,

il Presidente di Commissione; anzi, in questa sede mi consentirà di ringraziare il presidente Balboni perché si è ritrovato nella condizione di dover difendere il Regolamento: che un Ministro si esprima sulle modalità con cui è possibile intervenire sul complesso degli emendamenti, francamente a memoria non lo ricorda nessuno di noi. signor Presidente, che forse sia il caso che la maggioranza chiami un *timeout.* Non continuo con la lista delle gravi questioni che toccano la maggioranza, che la maggioranza conosce e che ci pare sempre più evidente non consentono una navigazione lucida di questo Governo.

Signor Presidente, anche per il Gruppo Movimento 5 Stelle ciò che sta accadendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza è fonte di grande preoccupazione, e non per una questione politica, ma per quel Piano è del Paese, e non del Governo o del Parlamento. È il Piano che deve rilanciare definitivamente il nostro Paese a livello economico rispetto alla digitalizzazione, alla transizione *green*

in carica del Governo Draghi e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza regna una confusione assoluta. Le Aule del Parlamento nulla sanno rispetto alle modifiche proposte; nulla sanno rispetto alla condivisione di queste modifiche nei consessi europei; nulla sanno sulle intenzioni del Governo rispetto all'utilizzo di tutte le risorse del Piano. Da parte di vari Ministri continuano a essere fatte dichiarazioni ambigue che si contraddicono una con l'altra. L'unica certezza L'unica certezza è che si è voluto spostare una cabina di regia, perdendo molti mesi, e che si è voluto cambiare tutte le strutture di missione di tutti i Ministeri per mettere le proprie persone in quei luoghi.

diciamo che il provvedimento e il Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono di questo Governo - tutto è iniziato col Governo Conte II, proseguito col Governo Draghi, in parte speriamo organizzato dal Governo Meloni e le conseguenze le vedranno altri Governi

Signor Presidente, colleghi, è per me un onore poter riferire all'Assemblea su un provvedimento che destina risorse per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma.

alla necessità di mantenere viva la memoria, soprattutto tra i più giovani, dell'orrore che ha investito anche il nostro Paese nel ventennio fascista con l'approvazione delle leggi razziali e che è culminato poi con la persecuzione e lo sterminio di decine di migliaia di ebrei italiani. Il nostro impegno principale - come ha ricordato anche il presidente Mattarella nella recente visita a Birkenau, accompagnato dalle sorelle Bucci sopravvissute alla Shoah, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere e il cui racconto ho potuto ascoltare dal vivo - deve essere proprio quello di evitare che tali orrori, in forme nuove e meno riconoscibili, possano ripetersi. Mi rispecchio totalmente nelle parole del presidente Mattarella che, alla studentessa che gli chiedeva cosa si prova a visitare quei luoghi emblematici, ha risposto nonostante si leggano tanti libri o guardino video, vedere dal vivo è tutta un'altra cosa, dà la misura dell'orrore e dell'immaginabile. Io stessa posso testimoniare quanto sia stato difficile trovarsi davanti agli occhi - solo per fare qualche esempio le protesi delle persone con disabilità ritenute vite non degne di essere vissute e uccise al loro arrivo nei campi di concentramento. In altre occasioni anche il Presidente della Repubblica ha avuto modo di ricordare a tutti noi che il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano. Sono un monito che dobbiamo tenere sempre a mente. Come in tante altre città, dove già esiste un museo della Shoah - a partire da Berlino, Gerusalemme, Milano, Varsavia, New York - era necessario che anche Roma, la capitale, dove pure la comunità ebraica ha saputo tenere vivo il tragico ricordo del rastrellamento del ghetto del 16 ottobre del 1943, si dotasse di un percorso museale dalla forte valenza educativa, non solo - appunto - per mantenere vivo il ricordo di un fatto storico, ma anche e soprattutto per generare quegli anticorpi che possano contrastare il virus sempre minaccioso del razzismo e dell'intolleranza. Credo che sia questo, in definitiva, lo spirito con cui oggi l'Assemblea deve approvare e licenziare il testo Passo quindi a illustrare brevemente il contenuto del provvedimento. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah costituita nel 2008 proprio dalla *mission* di dare impulso alla costruzione del Museo nazionale della Shoah a Roma e la partecipazione è finalizzata alla realizzazione del suddetto museo, nonché a contribuire a tenere viva la memoria della tragedia della Shoah. Il comma 2 affida la gestione del Museo alla Fondazione stessa. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce che la Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che prevede di fatto il coinvolgimento della Fondazione. Rispetto al testo presentato dal Governo è stata soppressa la disposizione che attribuiva al medesimo Ministero la programmazione delle attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 4 autorizza la spesa di 4 milioni per l'anno 2023, 3 milioni per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alle relative coperture finanziarie.

fra i miei primi atti in Consiglio dei ministri la richiesta di istituire un Museo della Shoah nella città di Roma. Chi ha seguito le cronache dei giornali sa che il mio primo atto, a pochi giorni dalla nomina a Ministro, è stato quello di recarmi in visita alla Sinagoga di Roma e il secondo atto è stato quello di recarmi presso quella che fu la casa di Benedetto Croce, che oggi ospita l'Istituto italiano per gli studi storici. Credo che con l'istituzione di questo Museo venga sanato un grave *vulnus* da parte della Repubblica, perché - come ha giustamente ricordato la relatrice - un museo che ci dia la memoria della Shoah esiste in tutte le grandi capitali occidentali e, quindi, è bene che ci sia anche in Italia. Lo ritengo pertanto un atto qualificante. Altre iniziative ci sono state, e ricordo il museo di Ferrara, ma il fatto che esista non significa che non ce ne possa essere un altro nella città di Roma: nella città di Roma: abbiamo assolutamente il dovere di coltivare la memoria di quella che è stata la Shoah, per la quale ritengo che ci sia stata un'unicità storica dell'orrore. Ringrazio il presidente Mario Venezia per il lavoro che ha fatto negli ultimi anni per tenere viva la memoria di questo evento e avrà al mio fianco tutto il sostegno, affinché la Fondazione possa prendere e gestire accuratamente il Museo. Ringrazio tutti gli amici della comunità ebraica, che vedo l'espressione il dovere della memoria, perché - come dice Benedetto Croce - la storia non è soltanto un fatto contemporaneo. Croce ci dice che la storia è una sorta di cassetta degli attrezzi, nella quale possiamo rinvenire gli elementi per interpretare il presente e magari proiettarci verso il futuro. Quindi, il dovere della memoria non è soltanto un fatto di rievocazione storica, ma è anche un qualcosa che deve generare gli anticorpi nella nello spirito di ciascuno di noi, affinché si mantenga alta la guardia verso ogni atto di antisemitismo. Fatemi dire solo una cosa: il Museo è stato a lungo teorizzato trent'anni si parlava nella città di Roma del Museo della Shoah. Noi con grande umiltà lo abbiamo fatto e vi ringrazio se vorrete votare a favore del provvedimento in

io non riesco a essere felice nel parlare di questo Museo, e non perché non sia d'accordo, ma perché la

e che potrebbe in qualunque momento riaccadere mi provoca davvero dolore, un dolore profondo, forse senza sensi di colpa. Non sono di quelli che si fanno carico delle colpe degli altri, ma certo in qualunque momento della storia piccola e grande della cosiddetta umanità quello che è accaduto anche prima della Shoah in sé non ha precedenti

e penso che la vita sia meravigliosa in ogni caso e vada difesa sempre, senza supponenza, senza violenza e con dolcezza. Ma certo quello che è accaduto nella Shoah non ha precedenti. Debbo dire un minimo di orgoglio - ma nessuno di noi si può appropriare in maniera quasi narcisistica del dolore collettivo degli altri - che qualche anno fa - in quel momento ero fuori dal Parlamento - con l'allora presidente della Camera Gianfranco Fini organizzai un convegno di riflessione assieme alla Comunità Papa Giovanni. Ricordo che facemmo una ricerca sui precedenti della Shoah, perché la macchina di morte e di umiliazione che ha scatenato quel periodo

C'è stato un tristissimo e orribile rodaggio per vedere come uccidere più persone possibili,

Debbo dire che in quella giornata dolce e terribile dicemmo quello che abbiamo sempre - ahimè - saputo, ossia che a rodare soprattutto l'efficienza dei forni crematori

accanto a loro e con loro, persone con disabilità, rom e persone con scelta sessuale per quei tempi diversa: un triste rogo di esperienze per far sì che si potessero uccidere sempre più persone, prima umiliate e poi date al fumo. Sono convinto che realtà - dire orribili è poco - come la Shoah sono uniche nella storia, ma non è detto che non si ripetano in tante, piccole terribili realtà. Non dobbiamo rimuoverci la coscienza; una parte di quello che è accaduto può riaccadere in maniera magari meno "organizzata", meno collettivizzata, ma sempre prevaricante, orribile e negante la diversità dell'altro. Se posso permettermi, senza nulla togliere al mondo ebraico,

si sbeffeggia magari una persona perché avente idee politiche diverse, si ripercorre almeno in parte la cosa peggiore, ossia la negazione dell'altro,

tutte le capitali europee hanno un museo della Shoah. Finalmente, con grande celerità e decisione, lo avremo anche da noi, a Roma, la città che ha vissuto

museo. Io dico meno male se ci sarà, ma non vogliamo un museo rappresentativo del passato. Vogliamo che sia presente ogni giorno con le scuole, con i cittadini del mondo, con i viandanti del mondo che spesso, soprattutto in questo periodo, non hanno una stella polare che gli dia la direzione giusta. Questo Museo può ricordare che può ancora accadere. Questo è fondamentale: ci deve mettere in guardia, perché - colleghi senatori quella che è stata la Shoah non deve essere fraintesa come restrizione in un periodo che si apre, si chiude e si mette nel Museo. L'intossicazione psicologica che ha condotto alla Shoah, magari in termini diversi, persino più orribili e più subdoli, può ancora accadere e allora sì, davvero, questo Museo può essere, se non un anticorpo decisivo, certamente un momento di prevenzione. È importante che sia

non mi stancherò mai di dire, a me stesso prima di tutto, che il virus dell'intolleranza, il virus ammalante, devastante del rifiuto della diversità del corpo, della razza, delle idee, delle scelte, delle appartenenze esiste sempre e può ucciderci nell'anima ogni giorno.

se morirà l'ultimo giusto - e l'ultimo giusto non è una persona eccezionale: è chiunque di noi, portatore di una piccola o grande diversità diversità - se verrà ucciso dal pregiudizio, prima ancora che dai forni crematori, l'umanità scomparirà, soffocherà, perché senza la libertà di espressione, che non si vede ma è come l'aria, moriremo

un pochino in colpa, perché si può fare di più e soddisfatti perché almeno adesso, per fortuna, qualcosa abbiamo fatto.

legge in esame, recante l'istituzione del Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah, già costituita nel luglio 2008 e avente sede a Roma, in via Portico d'Ottavia 29, è sicuramente un fatto positivo che, come ovvio, accogliamo favorevolmente. L'istituzione di un museo dedicato alla Shoah è infatti di fondamentale importanza, per molteplici ragioni. In primo luogo, tale museo rappresenterebbe un memoriale permanente per le vittime dell'Olocausto, onorando la loro memoria e preservando le testimonianze delle atrocità commesse durante quel periodo buio della storia umana. Un museo dedicato alla Shoah ha un ruolo educativo cruciale, offrendo agli individui la possibilità di conoscere in modo approfondito l'orrore dell'Olocausto. Attraverso mostre, documenti storici, fotografie e testimonianze dirette, il museo potrà contribuire a sensibilizzare le persone sulla necessità di combattere l'odio, la discriminazione e l'intolleranza. Inoltre, un museo di questo tipo può sicuramente svolgere un ruolo nel promuovere la comprensione interculturale e l'importanza del rispetto per le diversità. Attraverso l'analisi delle cause e delle conseguenze dell'Olocausto, il museo potrebbe potrebbe aiutare a prevenire il ripetersi di simili tragedie nel futuro e servirà altresì come centro di ricerca e studio, offrendo agli studiosi e agli storici un accesso diretto ai documenti e agli archivi relativi all'Olocausto. Questo contribuirà a garantire che l'evento sia accuratamente studiato, compreso e trasmesso alle future generazioni, oltre a rappresentare un vero investimento sulla memoria. investire sulla memoria come strumento di conoscenza, per non dimenticare e svelare i processi che condussero e rischiano di condurre ancora a un nuovo totale oblio della ragione. In realtà, la persecuzione degli ebrei ha radici lontane nel tempo, ma è soprattutto nel 1933 che assunse il carattere a noi noto, quando fu varata una legge che decretava la sterilizzazione coatta di ogni individuo "inadatto alla propagazione". La categoria degli inadatti si sarebbe estesa negli anni successivi, per comprendere criminali, comunisti, omosessuali, zingari, diversamente abili e, naturalmente, ebrei. Una legge del 1936 vietava il matrimonio e ogni rapporto sessuale tra tedeschi ed ebrei. Dal 1939, l'eutanasia di chi non meritava di vivere fu vista come una soluzione preferibile alla sterilizzazione: spendere per nutrire pazzi, carcerati, degenerati ed ebrei? Si avviò così la costruzione delle camere a gas e dei forni crematori. Le torture che tutti gli "inadatti" dovettero subire furono innumerevoli. Oggi, in molti Paesi del mondo, avviene una sistematica violazione dei diritti umani, tra cui la pratica della tortura. Le carte dei diritti e le legislazioni internazionali unanimemente la condannano. Se è però vero che la tortura è vietata, certamente non è impedita e in molti, troppi casi è ancora praticata. La memoria costituisce l'unico appello che il sopravvissuto Primo Levi rivolge all'umanità: il dovere di non dimenticare ciò che è stato. La sua lucida testimonianza non si prefigge di formulare capi d'accusa, né di aggiungere altri elementi a ciò che è ormai noto, ma di indagare in modo pacato alcuni aspetti dell'animo umano. Il timore di non essere creduti e la vergogna di rendere note le umiliazioni subite hanno per lungo tempo tenuto in carcere vittime e testimoni. Il dovere morale che l'esperienza dei *lager* impone è quello di spezzare la forza che la tirannide continua ad esercitare, anche molto tempo dopo che quelle prigioni sono state smantellate. La creazione di un museo dedicato alla Shoah sarà un impegno tangibile per la preservazione della memoria storica e della verità. Attraverso la commemorazione delle vittime e la narrazione delle loro storie, il museo potrebbe fungere da luogo di riflessione e di meditazione, incoraggiando un confronto critico con il passato. Inoltre, il museo potrebbe servire come punto di incontro e di dialogo, promuovendo la comprensione reciproca e la costruzione di legami di solidarietà. La sua presenza potrebbe contribuire a combattere l'antisemitismo e ad affrontare il negazionismo dell'Olocausto, offrendo una smentita visibile ai tentativi di distorcere la storia. Infine, permettetemi di dire che, da queste riflessioni e dall'istituzione di luoghi come questo, dovremmo saper cogliere elementi di positività, per migliorare il nostro presente. Per tornare ai giorni nostri e alle ferite che si riaprono in nuove, drammatiche rappresentazioni sociali di odio xenofobo, è necessario comprendere quanto la relativizzazione spinta delle differenze porti ad esiti paradossali di indifferenza le differenze altrui (a salvaguardia del proprio gusto e spazio di scelta), sulle quali bisognerebbe invece essere più profondi e su cui in quest'Aula abbiamo il dovere di riflettere, pensando anche alle conseguenze, anziché speculare ed enfatizzare, come qualcuno fa, innescando pericolosi rischi per la democrazia e per il bene comune.

È una legge giusta, quella che ci accingiamo a votare, ed è una legge che voteremo tutti insieme, nella convinzione che avere un museo della Shoah nella città di Roma sia un un giusto segno e sia un passaggio fondamentale di sottolineatura di un pezzo della nostra storia, che certamente non fa mai piacere ricordare e che - diciamoci la verità - noi italiani abbiamo tentato di rimuovere nei decenni, ma che resta una macchia indelebile nella storia del nostro Paese.

gli italiani di religione ebraica, erano cittadini di seconda categoria, anzi non erano cittadini; erano a loro precluse le professioni liberali ed era a loro precluso l'insegnamento. Non possiamo dimenticare le parole della nostra collega, la senatrice Liliana Segre, che proprio nella seduta inaugurale di questo Senato ci ha ricordato quando dovette lasciare la sua scuola elementare soltanto per la colpa di essere nata. Quelle leggi razziali produssero i loro effetti nel silenzio del Paese. Non si levò una voce per difendere gli insegnanti cacciati dalle scuole; non si levò una voce per difendere i bambini che, come la piccola Liliana, venivano buttati fuori dalle scuole; non si levò una voce

della Gestapo rastrellarono il ghetto di Roma, portando via donne, uomini, bambini e anziani, che praticamente tutti non tornarono più a casa. Noi abbiamo il dovere di ricordare. È un dovere che resta impresso nelle parole terribili terribili e spietate, giustamente spietate, di Primo Levi, che ci ammonisce sempre a ricordare quello che è stato. Io penso che dovremmo ricordarlo e farlo nostro, signor Ministro, perché spesso ci siamo detti che noi italiani eravamo brava gente, ma dietro questo nostro essere brava gente si sono nascoste cose terribili, che la nostra storia, come quella di molti altri Paesi, ha avuto soprattutto in quella fase, nella quale il nostro Paese ha strangolato il tentativo di democrazia liberale

oppositori e che cancellò la dignità di questo Parlamento. Qualcuno (Mussolini) nell'Aula di Montecitorio ricordò che avrebbe potuto trasformarla in un bivacco di manipoli. manipoli. E noi, che stiamo seduti in questo Parlamento, dobbiamo sempre ricordare che queste Aule hanno corso il rischio di essere trasformate, appunto, in un bivacco di manipoli e in un gruppo di persone che, minacciate dalla violenza fascista, erano tenute soltanto a dire di sì. Ecco, signor Ministro, io penso che questa sia una grande occasione non soltanto per continuare a ricordare quello che è stato, perché è evidentemente l'unica ricetta che abbiamo per evitare che che quello che è stato si ripeta, ma anche per fare un ragionamento su di noi, per appropriarci di questo pezzo di storia così doloroso, perché tutto ciò accadde in Italia. Certamente, come alcuni colleghi hanno già ricordato, le teorie antisemite erano più antiche, ricordo però che giornali come «La difesa della razza» erano stampati in questo nostro Paese; c'era proprio una sorta di gioco scientifico a descrivere descrivere i tratti somatici di quelle persone, che non potevano essere considerate umane. Vogliamo ricordare poi gli scritti che circolavano, come «I protocolli dei

Dobbiamo ricordare anche che di genocidi ne abbiamo visti tanti, ma chiunque abbia avuto l'occasione di visitare i campi di Auschwitz e Birkenau ha potuto vedere e toccare con mano quanto, in in nome di una ideologia politica che aveva deciso di individuare un capro espiatorio, si creò una vera e propria macchina dello sterminio, una macchina ingegneristica perfettamente oleata, che aveva come obiettivo quello di uccidere quante più persone possibile e di distruggere le tracce di quel genocidio e di quei corpi nel modo più

nel quale si possano consultare documenti o ripercorrere la tragica storia di quei giorni. Io credo che debba essere un'occasione per riflettere più in generale sulla dignità delle persone, sull'uguale diritto di tutte le minoranze a essere riconosciute davanti alla legge come uguali ai propri concittadini, che debba essere un pensiero costante a cosa significhi l'esistenza di cittadini,

capitale, precisamente in questa città. Grazie, signor Ministro. Presidente, colleghi, signor Ministro, diciamo subito che il Gruppo Forza Italia è certamente favorevole al disegno di legge in esame. È bene che preveda la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah, istituzione benemerita, costituita da circa quindici che ha sede in via del Portico d'Ottavia, cioè nel cuore del cosiddetto ghetto ebraico di Roma. Il Museo della Shoah è quindi il luogo per far conoscere a tutti cosa è veramente stato l'Olocausto e le assurde atrocità che lo hanno caratterizzato. Non ci sono parole, né pensieri sufficienti per poter comprendere ciò che non è comprensibile, ma il museo di Roma può e deve servire a creare una nuova coscienza in questa città, che è tra quelle con il maggior numero di turisti al mondo e che può aggiungere un ulteriore luogo di cultura ai tanti luoghi storici che ogni giorno vengono visitati. Deve essere aperto anche alle visite didattiche delle scuole: questo deve essere l'obiettivo, questo può e deve essere il percorso da seguire. Ciò si pone anche in continuità con quanto già fatto dal Senato in questa legislatura, in cui abbiamo approvato il disegno di legge sui viaggi della memoria degli studenti proprio nei luoghi in cui queste infamie dell'Olocausto furono perpetrate. Va ricordato che sono soci fondatori di questa fondazione l'Associazione figli della Shoah, la comunità ebraica, istituzioni come la Regione Lazio, Roma Capitale e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. La fondazione viene giustamente posta sotto la vigilanza e la guida del Ministero della cultura; viene anche prevista un'adeguata dotazione finanziaria, perché sia possibile realizzare e implementare il funzionamento del museo. Stiamo parlando di circa 10 milioni in tre anni. Il risultato è che viene valorizzato un ulteriore luogo di conservazione della memoria, che va ad affiancare il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara, creato ora nel luogo dove la comunità ebraica italiana segna la maggior presenza nella capitale. È già stato ricordato: purtroppo, però, è proprio da Roma che nel 1943 partì la deportazione nazista di oltre 1.000 ebrei romani, quindi anche in questo senso avrà un forte significato simbolico. Il testo con cui il Governo intende assumere la vigilanza della fondazione è stato ulteriormente migliorato dal lavoro della 7a Commissione, quindi anche per questo il Gruppo Forza Italia conferma il proprio voto favorevole. una svastica tatuata sul petto all'altezza del cuore, un fascio littorio sulla gamba destra, simbologia e frasi che richiamano alle Schutzstaffel (SS), al nazismo e al fascismo tatuate su tutto il corpo. Il 2 luglio è questa la scena che si è presentata agli occhi di molti turisti nella spiaggia di Cala Pisana a Lampedusa non ha lasciato indifferenti i presenti. Il primo ad esprimere il proprio disagio è stato un austriaco di trentasette anni, JaKob Brossman, scenografo e regista di documentari, noto per il film documentario «Lampedusa in winter». Brossman, fortemente provato, ha fermato sulla battigia l'individuo di origini romane, facendogli notare di risultare offensivo ai presenti e alla storia; dall'altra parte, la replica è stata prepotente e negazionista. In pochi minuti, però, il regista ha trovato il conforto nella reazione educata e compatta dei bagnanti presenti, che hanno dato manforte all'austriaco. Alla scena ho assistito personalmente, unitamente al collega Pietro Lorefice. In quei giorni, infatti, eravamo presenti sull'isola per approfondire i contorni di una vicenda drammatica, di cui, loro malgrado, sono protagonisti i vigili del fuoco di Lampedusa e per verificare la situazione critica dell'*hotspot,* sovraccaricato dall'arrivo in un solo giorno di 2.500 migranti. Tornando all'episodio poc'anzi descritto, quello che più mi ha turbata sono state due frasi con cui l'uomo ha ostentato disprezzo e noncuranza delle osservazioni di tutti noi: sto solo esprimendo la mia libertà di pensiero, siamo in democrazia e quindi posso dire quello che voglio. Poi ha aggiunto: voi siete ignoranti, non sapete cosa significa questo simbolo (indicando la svastica tatuata sul capezzolo). Tutto questo mentre le sue due figlie, tra i sei e i dieci anni, assistevano in silenzio alla scena. Riguardo alla prima frase, è stato inevitabile considerare che, se fino a pochi mesi fa queste esibizioni di supremazia della razza e neofascismo si consumavano prevalentemente nei raduni di estremisti e di nascosto, oggi sembra che questa gente non abbia più vergogna di niente, galvanizzata anche da chi ha sdoganato la nostalgia di teorie sulla sostituzione etnica, con la banalizzazione, la rivisitazione di pagine storiche e l'attacco ai diritti di chi non rientra, ad esempio, nei canoni della famiglia tradizionale. *(Applausi. Commenti)*. Riguardo alla seconda frase, mi sono limitata a ricordare a quell'individuo che quel simbolo rappresenta lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Avrei dovuto sicuramente fare di più: ad esempio, raccontare - confidando che ascoltassero soprattutto le sue due figlie - cosa è successo il 16 ottobre del 1943. Mi dispiace che i colleghi dai banchi della maggioranza, per suo tramite, Presidente, vogliano minimizzare evidentemente quello che purtroppo è un fatto accaduto, di cui sono testimone oculare; e mi sembrerebbe corretto non tanto nei miei riguardi, ma nei riguardi di tutti coloro che sono stati offesi dall'Olocausto prestare attenzione a quello che sto raccontando. Era un sabato, *shabbat*, il giorno di riposo per gli ebrei, l'occasione perfetta per un centinaio di SS al comando di Kappler che arrivarono nell'ex ghetto con i camion, con la svastica e le SS ben riconoscibili sulla loro divisa, proprio i simboli ostentati dall'individuo sulla spiaggia di Cala Pisana. Raggiunsero ad una ad una le abitazioni agli indirizzi forniti dall'ufficio fascista demografia e razza e bussarono alle porte, che non esitarono a sfondare in mancanza di una pronta risposta dall'interno. Impassibili e arroganti, lessero l'ordine perentorio dattiloscritto: "Dovete essere pronti in venti minuti, portare cibo per otto giorni, soldi e preziosi, con voi anche i malati. Nel campo dove vi porteranno c'è un'infermeria". Nello stesso tempo, con identico metodo, negli altri quartieri di Roma si procedeva alla caccia all'ebreo: uomini, donne, bambini, anziani, ammalati e perfino neonati, tutti deportati nei campi di sterminio, da cui solo in pochi tornarono. Il simbolo della svastica nell'immaginario collettivo dovrebbe essere legato a orrore e disgusto per queste e altre nefandezze di cui si è reso colpevole chi lo ostentava. Anche un solo individuo che ne ignori il peso nella storia è un colpo inferto alla memoria della Shoah, a quel patrimonio dell'umanità tributo alle vittime del genocidio degli ebrei d'Europa e dello sterminio di tutti coloro che per motivi politici o razziali fossero ritenuti inferiori, la memoria dei crimini di cui si resero responsabili il Governo nazista e i loro alleati fascisti nel corso del Secondo conflitto mondiale. Perché la memoria non solo venga preservata, ma soprattutto venga veicolata e si connetta attraverso più canali possibili a più soggetti possibili, come MoVimento 5 Stelle non possiamo che accogliere con estremo favore la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah. Ci auguriamo che questo passo definisca con chiarezza e senza fraintendimento alcuno le azioni concrete con cui il Ministero concorrerà a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e contribuirà a realizzare a Roma il Museo della Shoah. Ritorno all'episodio di Lampedusa - e concludo, Presidente, annunciando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle - per raccontare che, dopo l'acceso confronto, il nazifascista si è spostato dalla parte opposta della spiaggia e ha indossato la maglietta. Se non fosse stato solo e avesse trovato il conforto di altri sodali, forse l'epilogo sarebbe stato diverso, ma voglio credere che le parole di tutti i presenti abbiano potuto instillare un minimo dubbio nelle sue convinzioni e confido ancora di più che in futuro le sue figlie, una volta che sarà realizzato, possano invitare il loro padre a visitare il Museo della Shoah per fargli conoscere cosa sono stati l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato. *(Applausi)*.

l'istituzione del Museo della Shoah è un'importante occasione per riflettere sugli accadimenti di un doloroso passato e, al tempo stesso, consolidare le basi e attivarsi perché nel presente e nel futuro le cause che generarono la Shoah non si ripresentino mai più. Ricordare e trasmettere la memoria è un impegno arduo, soprattutto in una società immersa nel presente e dominata dalla velocità. Si avverte sempre più l'esigenza di non restare su un argomento così drammatico, prigionieri di parole e di modalità di trasmissione che appaiono paradossalmente necessarie, ma al tempo stesso non del tutto efficaci, quando ci si trova di fronte al compito non facile di raccontare ai giovani e ai giovanissimi gli errori e le mostruosità di cui gli esseri umani sono stati capaci. Questo passato è spesso percepito da loro come distante e poco decifrabile, ma è fondamentale che la comunità si assuma il carico di trasmettere e mantenere viva la memoria, perché questa è in realtà indispensabile per orientarsi nel mondo e e implica scelte decisive tanto per l'oggi, quanto e soprattutto per il domani. I testimoni diretti della tragedia inevitabilmente tendono a scomparire e c'è il rischio che una parte crescente dell'opinione pubblica consideri l'Olocausto come un evento lontano che appartiene alla storia e al quale l'attualità ha pochi rimandi perché si ritiene che su di essa incidano problematiche profondamente diverse. Il riconoscimento della memoria e la condanna, apparentemente unanimi, a un esame più attento risultano fragili, insidiati non tanto dal revisionismo o dal negazionismo, quanto piuttosto dal male sottile dell'indifferenza. Perciò, fra coloro che questa memoria vogliono custodire e vogliono farne discrimine, affiora il dubbio che negli anni la questione non sia stata sempre proposta nella maniera più efficace, stimolando la ricerca di diverse modalità narrative, soprattutto per affrontare la questione nelle scuole e tra i giovani. Le occasioni dedicate alla memoria sono state peraltro anche diversificate: sono numerose quelle affidate agli strumenti della creatività e dell'arte, in particolare cinematografica. Eppure, le campagne sulla memoria, anche se utili, non hanno sempre avuto l'effetto desiderato. Nei giovani può sorgere l'impressione che il tutto si risolva in una narrazione retorica, lontana dalle problematiche della società moderna. ha quindi bisogno, quasi l'urgenza, di coniugarsi con i nuovi linguaggi e con i nuovi mezzi di comunicazione, ma soprattutto di indicare nel tempo attuale ricorrenze e similitudini, senza appiattirle e - illuminandole - illuminare se stessa. La memoria dell'Olocausto può infatti essere resa più comprensibile con riferimenti alle diverse, ma comunque atroci discriminazioni, ingiustizie e violazioni dei diritti umani che sono purtroppo presenti in molte aree del mondo. Quell'odio e quell'idea di superiorità razziale, culturale e ideologica che portarono al genocidio di un intero popolo e che costruirono l'orrore di Auschwitz sono ancora vivi, anche se non si ripetono nelle stesse forme e non agitano uguali parole d'ordine. Negli ultimi anni, si è purtroppo registrato un aumento di fenomeni ed episodi spesso apertamente antisemiti, ad esempio nel mondo dello sport. Qualche mese fa, la FIFA ha dovuto revocare all'Indonesia l'organizzazione dei mondiali di calcio *under* venti e spostarla in Argentina, perché la stessa nazionale indonesiana e quella irachena - pensate un po' si rifiutavano di scendere in campo contro la rappresentanza di Israele. Vergogna, vergogna, vergogna! È anche per tutto questo e con le finalità che ho provato a indicare che considero veramente lodevole l'iniziativa di istituire a Roma il Museo della Shoah. Oggi abbiamo la piena consapevolezza che i musei, in quanto strumento di salvaguardia del patrimonio culturale, svolgono nella società un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo socioculturale e contribuiscono, in definitiva, allo sviluppo sociale e umano. dotandosi di un suo specifico Museo della Shoah, l'Italia e la città di Roma faranno un ulteriore fondamentale passo in avanti nel consolidamento del proprio ruolo di faro di libertà e di rispetto dei diritti umani. È per tutto questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. è con una certa emozione che, a nome del Gruppo Partito Democratico, dichiaro il voto favorevole su questo importante disegno di legge di iniziativa governativa che oggi siamo chiamati a votare e che abbiamo discusso e licenziato all'unanimità in 7a Commissione. Il disegno di legge in esame riconosce infatti l'importanza della costruzione nella nostra capitale di un Museo della Shoah. Con questo testo - lo hanno detto tutti - il Ministero partecipa alla Fondazione Museo della Shoah costituita nel 2008

ha fatto suo. Nei prossimi giorni saranno consegnati i cantieri e inizieranno i lavori a Villa Torlonia. Nel 2005 il sindaco Walter Veltroni lo rese un progetto dell'amministrazione capitolina, ma già da tempo, da prima del 2005, si ragionava di collocare nell'area intorno a Villa Torlonia un museo dedicato alla Shoah. Con Veltroni, dunque, il progetto prese corpo come progetto dell'amministrazione. Erano anni in cui Roma si presentava sulla scena come una città che voleva essere protagonista della cultura e un punto di riferimento. Erano anche gli anni in cui si affermava la religione civica della memoria, che si andava rafforzando e strutturando. Iniziava i viaggi della memoria, con la comunità e con l'amministrazione, la didattica della Shoah e la formazione degli insegnanti. Un museo nella capitale dedicato alla Shoah in Italia nasce per non dimenticare prima di tutto le responsabilità italiane nel genocidio degli ebrei. Ecco l'importanza della collocazione in quel quadrante di città dove Mussolini aveva posto la sua residenza. Acquistata l'area, vi furono poi varie vicissitudini, ma non starò a ripercorrere questa lunga storia, che oggi finalmente sembra vedere una fine. Nacque allora la fondazione del museo ad opera del comitato promotore, per dare impulso a questa costruzione. Oggi con questo finanziamento finalmente si ridà corpo e concretezza a un progetto firmato dagli architetti Luca Zevi e Giorgio Tamburini, che affiancherà e completerà i musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città europee e del mondo e - si badi bene - si affiancherà alla fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, non non per sovrapporvi. L'Italia ha un museo dedicato alla Shoah e quello a Roma non intende sovrapporsi, come non vuole farlo con altri luoghi molto importanti e significativi della memoria (penso al Memoriale della Shoah di Milano). Anzi, il Museo della Shoah di Roma potrà essere il nodo di una rete di istituzioni dedicate e non sfuggono l'importanza e il valore di avere nella capitale un simile luogo - da qui l'importanza anche della scelta del Ministero

come spiega Zevi: «perché in qualche modo la Shoah è un suicidio culturale e civile dell'Europa». Il progetto di sterminio degli ebrei e di altre minoranze è un suicidio perché nell'attaccare gli ebrei e tutte le minoranze (come i rom e i sinti), e i portatori di handicap e cittadini affetti da malattie mentali, è negare i valori europei. È una scatola nera sospesa sopra le nostre teste, per dire che è un problema con cui non possiamo fare i conti troppo rapidamente, né che sarà facile elaborarlo». Il Museo sarà il luogo che permetterà di conoscere che cosa sono state le l'atrocità che hanno caratterizzato l'Olocausto. Visitare un museo può essere un viaggio emozionante, un'esperienza formativa che mette in contatto con la propria civiltà. Nell'idea del museo c'è l'interesse per la trasmissione alle generazioni future di un lascito culturale e la costruzione di un patrimonio condiviso da rendere accessibile al pubblico, affinché ciascuno ne faccia esperienza. Questo farne esperienza ognuno singolarmente, ma in una dimensione condivisa, è ciò che fa nascere il sentimento di appartenenza a una storia: i musei sono un'infrastruttura della conoscenza, resi tali dal carattere permanente che hanno. Ecco perché è così importante dargli carattere permanente, dedicando un museo alla Shoah, il più grande crimine dell'umanità perché quella ferita rimanga segno della nostra storia, della memoria di ognuna e di ognuno, oltre la sopravvivenza dei testimoni. Sui mattoni della scatola nera ci saranno i nomi delle e degli ebrei romani vittime della Shoah, per guardare negli occhi gli orrori, perché Roma è stata atrocemente ferita, come ricorda anche la relazione introduttiva al disegno di legge. Questa città è sede di una delle più antiche comunità ebraiche. Ha una sua giornata della memoria, il 16 ottobre del 1943, e ci avviciniamo all'ottantesimo anniversario: 1.259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambine bambine e bambini di religione ebraica vennero prelevati dalla loro casa per essere deportati ad Auschwitz. Poche settimane dopo l'armistizio dell'8 settembre, la politica di deportazione si abbatté sul nostro Paese e la prima grande deportazione cominciò a Roma, alle prime luci dell'alba, nell'area del cosiddetto ghetto, dove molti avevano continuato ad abitare anche dopo la fine della ghettizzazione forzata, perché Roma capitale significava anche la fine della ghettizzazione forzata, va ricordato. Tutta Roma, però, era stata divisa in 26 zone d'azione. Alle dipendenze di Kappler e Dannecker, già responsabile delle deportazioni antiebraiche in Francia, si muovevano 365 uomini appartenenti alle truppe di occupazione tedesche, coadiuvati dalla questura di Roma e dalla polizia fascista. Tutte le persone vennero caricate a forza sui camion e portate a via della Lungara, a poca distanza da San Pietro. Qui furono fatte fermare: vennero liberate alcune persone non ebree e ripartirono il lunedì 18 ottobre dalla stazione Tiburtina, su 18 carri bestiame con destinazione Auschwitz. cento di loro venne ucciso immediatamente con il gas, appena arrivati. 147 uomini e 47 donne furono arruolati. Si salvarono in 16: una donna, Settimia Spizzichino, e 15 uomini. Nessun bambino è tornato indietro. Di tanti di questi bambine e bambini, l'archivio della Croce Rossa di Bad Arolsen ha restituito volti e nomi. Nel 2012 la Provincia di Roma ne fece una pubblicazione, curata da Umberto Gentiloni e Stefano Palermo, che per me, e credo per chiunque abbia potuto sfogliarla - c'è qui Riccardo Pacifici, che ne ha curato anche l'introduzione *(Applausi)* - è difficile dimenticare ed è giusto che sia così. Deportati e uccisi per la sola ragione di essere nati: nessun negazionismo potrà cancellare quello che è stato e contro ogni negazionismo dobbiamo rendere il nostro impegno e rinnovarlo ogni giorno. In tutta Italia, tra il 1943 e il 1945, gli ebrei deportati furono 7.495 (quelli romani 2.091). Una tragedia mostruosa è stata possibile, l'umanità ha perso se stessa: questa consapevolezza va diffusa e fatta conoscere per non dimenticare mai; va rinnovata di fronte al neonazismo dei nostri tempi e a questo serve un museo, che è un luogo vivo, attivo e partecipato. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Signor Presidente, signor ministro Sangiuliano, sono lieta della sua presenza, perché è alla cronaca il suo impegno fruttuoso, che ci ha permesso di arrivare oggi qui in Aula. Onorevoli colleghi, permettetemi di salutare in tribuna il neopresidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun *(Applausi)*, assieme ad altri consiglieri, ed anche il presidente della Fondazione del Museo della Shoah di Roma, Mario Venezia. Giunge oggi in Aula il disegno di legge di iniziativa del Governo per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. È una data importante, direi storica, Presidente, perché è da troppi anni che, nell'attesa della sua costruzione nella capitale, vi era la necessità di un sostegno significativo del Governo nazionale. Oggi è con orgoglio che possiamo prendere in mano questa iniziativa. La verità è è che, dopo Governi non eletti dal popolo, è il Governo Meloni, che gli italiani hanno scelto democraticamente, a poter finalmente realizzare il Museo della Shoah Sono fatti, signor Presidente, e non sono vane parole. È un patrimonio che deve unire e non dividere, nel rispetto di coloro che sono sopravvissuti, come la cara senatrice Liliana Segre, a cui mando un caloroso saluto *(Applausi)*, e di uomini e donne ancora oggi tra noi, come Sami Modiano e le sorelle Andra e Tatiana Bucci, a cui rivolgiamo, noi tutti, un forte abbraccio *(Applausi)*. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno testimoniato e non sono più fra noi e a coloro che dai campi di sterminio nazifascisti non sono più tornati. Il 27 gennaio 2004, con grande slancio, venne realizzata la partita della memoria, allo stadio Olimpico, un evento nato da una visione di Riccardo Pacifici, qui presente, a cui rivolgo i saluti. Riuscirono a portare, per quell'evento, Elie Wiesel: lo scopo era quello di mettere in agenda la realizzazione di un Museo della Shoah a Roma. Oggi, più che mai, con l'inesorabile scomparsa dei sopravvissuti allo sterminio, sentiamo la necessità e il dovere di agire, non solo perché i giovani hanno la necessità di farsi carico dell'essere a loro volta sentinelle della memoria, ma perché è triste e grave dover evidenziare che nel nostro Parlamento ci sono ancora linguaggi inaccettabili, come ciò di cui siamo stati purtroppo testimoni. un fatto che è accaduto nei giorni scorsi alla Camera dei deputati. A tal riguardo, attraverso lei, signor Presidente, mi rivolgo alla collega e senatrice Bevilacqua,

«Quando leggo decreto lavoro, mi viene da pensare alla frase sul portone di Auschwitz: "Il lavoro rende liberi"». Pensavo che non si potesse arrivare mai a questo punto *(Applausi)*. Pensavo che un paragone di questo tipo non si potesse mai fare. Pensavo fosse una *fake news*, una notizia falsa, ed invece no. Si è poi scusata, ma questo testimonia che abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere, insieme ed uniti. È bene che quella deputata ricordi quali fossero le condizioni di vita, o meglio come si moriva, in campi come quello di Auschwitz e Birkenau. È un richiamo che dobbiamo ad ogni singolo cittadino che voglia fare paragoni futuri inaccettabili. In quei campi gli uomini e, soprattutto, le donne perdevano la loro identità, venivano marchiati come bestie e considerati pezzi. Signor presidente, i bambini venivano strappati dai seni materni e alcuni usati come tiro al bersaglio, lanciati in aria davanti ai loro genitori. Tutto prima che, poi, ognuno di loro trovasse la fine delle sofferenze nelle camere a gas e nei forni crematori. Le abbiamo sentite tutti le parole della senatrice Liliana Segre, quando con sofferenza ci ha donato il suo racconto. Lì non c'era umanità, lì c'era l'inferno. Vede, signor Presidente, sono orgogliosa che questo Governo possa essere promotore di un'iniziativa come questa. E questa destra, che nella campagna elettorale veniva demonizzata e raccontata come impresentabile, le cose le sta facendo ed ora sono in imbarazzo loro, perché si trovano davanti al fatto nuovo che non avevano messo in conto, ovvero che il Governo della destra le cose le dice e le fa, e anche bene. Presidente, questo Governo, con a capo Giorgia Meloni, fa solo quello che è negli interessi degli italiani. Si sono stupiti del decreto anti-*rave*. Ma volevano la nostra Nazione invasa, da tutta Europa, per i *rave* abusivi? Si sono stupiti delle politiche sul lavoro, ma intanto il PIL cresce e l'occupazione sale, mentre in Europa siamo finalmente tornati protagonisti. Con il Governo Meloni tornano le scelte e vede, signor Presidente, tra queste scelte c'è anche quella di fare il Museo della Shoah, come quello della memoria delle Foibe, perché abbiamo il dovere di consegnare alle generazioni future la condivisione di questa memoria, che ha lacerato tutti noi italiani in un lutto che per troppo tempo è stato elaborato solo da una parte della nostra Nazione, in ossequio alla narrazione post-comunista che ha cercato al riguardo l'oblio. Nessuno deve avere paura della verità. Le dittature, tutte le dittature, falsano la storia, manipolando la memoria nel tentativo di imporre la verità di Stato. Queste parole non sono le mie, signori; sono del presidente della Repubblica Mattarella, e le ha pronunciate lo scorso febbraio. Già, la verità, signor Presidente, quella che spesso una parte politica omette; dittature che oggi, in nome del fondamentalismo islamico, vogliono imporre la loro visione della società nelle democrazie occidentali, privando *in primis* a noi donne ruoli che ci siamo conquistate in decenni di battaglie. *(Applausi)*. Un pericolo che trova proseliti in Europa ed in Africa, a danno dei cittadini colpevoli solo di essere cristiani od ebrei. Dopo l'inchiesta giornalistica di un quotidiano nazionale dei giorni scorsi (questa però è stata ignorata dalle opposizioni, non gli piaceva), è stato evidenziato come l'associazione, di cui è presidente Muhammad Hannoun, finanzierebbe Hamas, definita dall'Unione europea organizzazione terroristica. Se fosse vero, sarebbe gravissimo. Nonostante questo, la deputata onorevole Laura Boldrini ha detto di non ricordare se l'incontro con il presidente di quella associazione ci fosse stato o meno. siamo così gentili da rinfrescarle noi la memoria, invitandola a rivedere tutto quello che riporta la Rete dell'avvenimento, foto comprese. Concludendo, signor Presidente, oggi, anche con questo voto, Fratelli d'Italia conferma la sua coerenza. Quindi annuncio il voto favorevole alla realizzazione del Museo della Shoah di Roma e a tutte le altre iniziative che andranno nella direzione della testimonianza della verità. Ringrazio il Governo e ringrazio il ministro dei beni culturali Sangiuliano per gli sforzi profusi al riguardo, che rendono onore a tutti gli italiani.

Il Museo che renderà viva la memoria della Shoah è anche significativo che sia unito a un fatto culturale, perché è sotto la vigilanza del Ministero della cultura, e credo che sia un

con il seguente titolo: *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni

L'Atto Senato 693 reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria agli atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte. Vorrei soffermarmi solo ed esclusivamente su due aspetti. Il primo aspetto è volto a chiederci se effettivamente era necessario intervenire in questa materia. La risposta, a mio avviso, è positiva; c'era necessità di intervenire perché gli atti di vandalismo ai quali stiamo assistendo non sembrano affatto

La seconda riflessione riguarda le caratteristiche del disegno di legge al nostro esame che, anche grazie all'approfondito esame da parte della Commissione giustizia, introduce un sistema diretto ad includere una risposta sanzionatoria per tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici. La scelta è stata quella di contrastare questi atti di intollerabile vandalismo attraverso la previsione di sanzioni amministrative

Si è fatta però un'ulteriore scelta per mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio e, per rispettare la necessaria proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate in conformità ai recenti e ben noti orientamenti della giurisprudenza sovranazionale interna in relazione al cosiddetto *ne bis in idem*, al comma 7 dell'articolo 1 abbiamo previsto che l'autorità, sia essa giudiziaria o amministrativa, che si pronuncia per la seconda volta debba necessariamente tenere conto, al momento dell'erogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già erogate. Per quanto riguarda l'esame degli articoli, c'è un testo scritto che, come già detto,

il contrasto delle attività di deturpamento delle opere d'arte, l'ho fatto perché, come tutte le disposizioni legislative e repressive, nessuno vorrebbe mai farle, tenendo tutti alla massima libertà dell'individuo, ma ci sono dei momenti in cui il contratto sociale ci impone di agire se certi comportamenti eccedono la normale tolleranza. Come giustamente ha richiamato la senatrice Bongiorno, la prima obiezione che normalmente veniva fatta in merito ad un intervento legislativo su questa materia era data dal fatto che già vi fosse nel codice penale la punizione per chi imbratta o per devasta beni artistici. Bene, però c'è un piccolo problema;

o, in generale, di imbrattamento asseritamente simbolico continuavano. Io non voglio discutere le motivazioni, perché tante volte cercando di parlare con questi imbrattatori viene fuori che lo fanno per un buon motivo.

ce ne sono pochissime, si contano sulle dita delle mani, perché il bronzo era prezioso e a un certo punto, in momenti meno elevati della cultura e della storia dell'uomo, si è pensato che ci potessero essere degli utilizzi migliori per quel bronzo. modo, dei capolavori assoluti della scultura, che sono ancora alla base del nostro stesso sentire (perché la scultura greca è quella da cui poi discende tutto il nostro senso del bello, anche quello attuale), sono finiti in qualche fornace per creare qualche prosaica armatura o spada o cannone o altri strumenti magari di morte o di distruzione. noi abbiamo il monumento meglio preservato dell'antichità romana, il Pantheon; ciononostante è ben noto che in passato, per degli usi non particolarmente migliorativi rispetto a quello attuale, i giunti di bronzo delle travi del Pantheon vennero utilizzati per fare cannoni da mettere a Castel Sant'Angelo. Si pensi anche alle varie conquiste arabe in zone del mondo dove, in omaggio all'obbligo di non avere la rappresentazione di Dio, tanta arte sacra è stata cancellata, annullata, stuprata, graffiata; quante situazioni abbiamo visto in cui, per celebrare cadute di imperi, di regimi o qualcosa del genere, si è ben pensato di abbattere opere d'arte dal valore magari inestimabile. successo semplicemente per motivi futili: periodi in cui il viaggiatore pensava che fosse intelligente (e ogni tanto qualche cretino c'è ancora)

so solo che un'opera d'arte è un patrimonio dell'umanità; l'opera d'arte ci viene consegnata per essere tramandata in futuro, quindi noi siamo custodi dell'opera d'arte: non è mia, né di un altro, né di nessuno; l'opera d'arte è dell'umanità e come tale abbiamo il dovere di custodirla integra il più possibile. In certi casi ci sono stati dei miracoli, perché è ovvio che le guerre sono state per tanto tempo una delle più grandi occasioni di distruzione delle opere d'arte. Si pensi a un capolavoro come «L'ultima cena»,

veramente miracoloso, con dei sacchetti di sabbia temendo che gli eventi bellici avrebbero potuto danneggiarla. Guarda caso, una bomba cadde proprio nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie e soltanto il fatto che i frati, veramente illuminati in quel caso probabilmente dallo Spirito Santo, occultare e di proteggere il capolavoro di Leonardo con dei sacchi di sabbia ci consente oggi di avere la fortuna di poterla osservare ancora.

non andiamo tanto lontano, perché innanzitutto dovremmo dare corso all'idea che se c'è un vetro si può utilizzare quell'opera d'arte come un muro da graffiti

c'è stata una certa inerzia, ma fortunatamente ci si è accorti dopo un po' che le cose stavano andando fuori controllo, quindi si è aggiunta un'altra proposta di legge da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia e alla fine è stato emanato il testo del ministro Sangiuliano.

- siamo tra l'altro in periodo di riforma della giustizia - che magari qualche magistrato eccessivamente interpretante della legge dicesse che effettivamente non si danneggiava l'opera d'arte, ma soltanto il vetro e potesse utilizzare questa scappatoia per far sì che diventasse utile, consentito o possibile andare a imbrattare tutti i quadri di una mostra, oltretutto impedendo anche ai cittadini di vederla. Sempre qui a Roma, «Il seminatore» di Van Gogh, in prestito da un altro museo,

comunque veramente contento che questa proposta sia finalmente arrivata in Aula dopo tanti mesi, perché penso che non stiamo facendo un dispetto a chi protesta, bensì un servizio a chi verrà dopo di noi, dimostrando che abbiamo cura dei beni che i nostri padri ci hanno lasciato.

Signor Presidente, intervengo sul merito del disegno di legge, ma poi concluderò anche sull'ordine dei lavori. Sul merito, abbiamo affrontato questo provvedimento in Commissione con spirito laico, aperti alla discussione, anche se devo dire che quello che è arrivato e anche quello che è uscito dalla Commissione è un provvedimento molto pasticciato dal punto di vista tecnico-giuridico.

colpisce, imbratta e deteriora i beni culturali del nostro Paese. Siamo tanto favorevoli a una sanzione adeguata che la legge di riordino sui reati contro il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese porta il nome di due nostri ministri, Dario Franceschini e Andrea Orlando *(Applausi)*, che nella scorsa legislatura hanno portato a conclusione una legge di riordino che ha allineato il nostro Paese ai sistemi giuridici più adeguati a contrastare questi fenomeni. Quando la Presidente si è posta la domanda, anche prima nella sua introduzione, se fosse necessario questo intervento normativo e si è data una risposta affermativa, la nostra valutazione è che la considerazione della Presidente sia molto discutibile, se non altro per il fatto che - come lei stessa ha ricordato

Non c'era e non c'è oggi un vuoto normativo nel nostro Paese per sanzionare queste condotte, tant'è vero che il disegno di legge, lungi dall'introdurre nuove condotte non previste dall'ordinamento giuridico italiano, si limita a introdurre due nuove fattispecie, che sono identiche a quelle già previste dalla legge Orlando-Franceschini, che però punisce a titolo di sanzione amministrativa. Il disegno di legge riscrive due fattispecie, che tutelano appunto i beni culturali dal deterioramento e dall'imbrattamento, uguali e identiche a come sono scritte nel codice penale, semplicemente introducendo per quel tipo di condotta, oltre alla sanzione penale prevista dal codice penale, anche una sanzione amministrativa. Noi abbiamo fatto audizioni, nel corso dell'istruttoria in Commissione, di professori universitari che ci hanno spiegato che questo modo di legiferare è molto discutibile e, anzi, potrebbe addirittura profilare qualche rischio di incostituzionalità, perché se una stessa condotta è punita sia con una sanzione amministrativa, sia con una sanzione penale, il rischio è quello di una sovrapposizione di sanzioni e di punizioni che può creare un cortocircuito nell'ordinamento.

il quadro della legge Franceschini-Orlando, introducendo una fattispecie particolare - che oggi non è prevista - che è quella dell'imbrattamento dei beni strumentali alla tutela dei beni culturali, cioè le teche e i siti dove sono protetti e conservati i beni culturali: tutti quei beni che sono funzionali alla conservazione e alla tutela dei beni culturali e che oggi non sono esattamente coperti dalle sanzioni previste dal codice penale. Questo nostro suggerimento, in realtà, è stato accolto, perché, nel corso dell'istruttoria e poi dell'approvazione degli emendamenti, è stato aggiunto un articolo in particolare che completa l'ordinamento sotto questo profilo. Per questo particolare aspetto siamo anche d'accordo, ma il punto è che la parte principale di questo provvedimento è semplicemente una duplicazione di sanzioni che già oggi sono previste, per condotte già previste e già punite dal codice penale, con sanzioni amministrative e con quei profili di criticità che prima ricordavo. Abbiamo presentato degli emendamenti sia in Commissione sia per l'Assemblea che cercano di contribuire a un miglioramento del provvedimento, intanto riducendo le sanzioni amministrative, che secondo noi sono smisurate anche tenendo conto dei criteri e dei principi di proporzionalità che devono giustificarne la misura. Sono sanzioni molto più elevate delle multe previste dalla sanzione penale e che non sono proporzionate a sanzioni analoghe per fattispecie con analogo disvalore nel nostro ordinamento.

non è che introduciamo una sanzione amministrativa perché oggi chi imbratta, chi deteriora, chi distrugge non sia tenuto a pagare: si paga sempre, perché c'è comunque il risarcimento del danno ai sensi dei principi civilistici.

abbiamo presentato degli emendamenti finalizzati ad abrogare l'articolo 1, che riproduce esattamente le condotte previste dal codice penale, duplicando una sanzione in modo secondo noi del tutto irragionevole.

nel caso in cui chi ha messo in atto la condotta ripristini lo stato dei luoghi,

Questi emendamenti li abbiamo offerti alla Commissione, che li ha respinti, per cui li ripresentiamo alla discussione dell'Assemblea sperando che possano essere accolti per migliorare un provvedimento che così com'è non ci piace. Concludo il mio intervento ricordando che oggi in Commissione i commissari del Partito Democratico sono usciti dall'aula quando è entrato il sottosegretario Delmastro

aspettando dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove delle scuse per le frasi che ha pronunciato successivamente ai noti episodi per i quali poi è stato anche indagato;

l'ex capogruppo alla Camera Serracchiani, l'ex responsabile giustizia del PD Verini, l'ex ministro della giustizia Orlando e un altro deputato che era con loro in visita a Cospito di essere andati a fare un inchino ai mafiosi. *(Commenti).* Ha quindi accusato i membri del Partito Democratico di essere dei mafiosi

In assenza di queste scuse, siamo usciti e continueremo a uscire dall'Aula della Commissione, e usciremo anche da quest'Aula nel momento in cui il sottosegretario Delmastro Delle Vedove prenderà la parola.

tutta la nostra totale vicinanza al sottosegretario Delmastro che è presente in Aula, quindi sono ben felice di queste interruzioni, per una volta. Venendo invece al motivo per cui ho chiesto di intervenire, nessuno pensava o ha pensato che

Penso però che il legislatore, quindi noi in questo caso, più persone, più senatori e anche il Governo, abbiano l'obbligo di stare attenti ai tempi che cambiano e di stare attenti anche alle modalità con cui chi deturpa, imbrattata e danneggia i monumenti lo fa. In passato, sinceramente, non avevamo mai visto casi in cui per protestare contro qualcosa, si imbrattava o si danneggiava un monumento. Abbiamo visto pazzi squinternati, gente senza cervello, ultras di qualche squadra di calcio, innamorati che perdono la testa e scrivono sui monumenti, persone che in corteo imbrattavano senza neanche saperlo. invece noi abbiamo dovuto vivere e affrontare una questione differente: esiste oggi chi deliberatamente imbratta, deturpa un monumento per protestare,

è la prova di una sensibilità comune secondo la quale questo modo di comportarsi non è gradito e non va bene. Poi ci sono i tecnicismi, c'è chi sostiene che il sommare la sanzione amministrativa alla sanzione penale non sia corretto, sia incostituzionale, politicamente, perché oltre che essere legislatori facciamo anche politica, penso che fosse e sia oggi necessario dire che gli italiani sono stufi di chi deturpa e imbratta i monumenti per affermare un concetto. È una sorta di terrorismo ideologico che impone a chi non è d'accordo comunque di vedere per più o meno tempo un monumento deturpato o imbrattato. È un danno all'immagine che

verso condotte che, è vero, rimangono le stesse, perché non c'è un modo diverso di imbrattare o deturpare un monumento, se non quello dell'azione manuale sul o contro il monumento. Mi sarebbe sembrato particolare che nella normativa si inquadrasse una nuova condotta, quindi, correttamente e giustamente, si decide di sanzionare anche dal punto di vista amministrativo un comportamento che non è tollerabile.

sui "ma" che si mettono davanti a questa norma, che invece ha colto, in senso molto positivo, il pensiero comune degli italiani, che dicono basta a un comportamento che non solo

relativamente alla fattispecie del deturpamento o dell'imbrattamento dei beni culturali e paesaggistici, al fine di offrire una opportuna risposta a quanto previsto dal disegno di legge governativo. Facendo seguito a quanto detto anche dal senatore Berrino, l'introduzione di un'ulteriore sanzione, in questo caso amministrativa, volta a punire la medesima condotta rispetto a quella già prevista dal secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, renderebbe irragionevole, irragionevole, maggiormente afflittivo e forse sproporzionato, e quindi incostituzionale, il trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo*. Essa predispone un doppio regime sanzionatorio che, andando a colpire sia per via amministrativa che penale le medesime condotte, si porrebbe in contrasto col principio *ne bis in idem*, allontanandosi da quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria. Il bilanciamento previsto dal comma 7 dell'articolo 1 non sembra sufficiente al fine di un'esclusione di eventuali giudizi di costituzionalità, che potrebbero e dovrebbero interessare la norma qualora fosse approvata *sic et simpliciter*. Infatti, il codice penale già prevede un sistema punitivo adeguato, all'articolo 518-*duodecies* del codice penale. Il disegno di legge governativo a ciò aggiunge anche una sanzione amministrativa. europea per i diritti dell'uomo (CEDU) ha da ultimo ritenuto il *ne bis in idem* compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio, quindi penale e amministrativo, in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti, nonché nei casi in cui sia assicurata la proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate, al fine di scongiurare un'eccessiva severità, e qualora i due procedimenti, per quanto non conseguenziali, non lascino il soggetto in un perdurante stato di incertezza processuale, protraendo eccessivamente i tempi di definizione. La normativa, quindi, si troverebbe disallineata rispetto a tale pronuncia, su diverse questioni, è relativa alle tempistiche di espressione dei provvedimenti conclusivi di diversi procedimenti. È infatti chiaro che il procedimento amministrativo sarà concluso nel giro di un breve periodo dal compimento del fatto, anche perché risiede proprio su tale questione la logica dell'intervento governativo. stesso discorso, ovviamente, non può essere fatto per quello penale, visti i tempi di definizione dei giudizi. Va da sé, quindi, che il soggetto sarà lasciato in un perdurante stato di incertezza processuale. Unitamente a ciò, vi è da considerare che un trattamento così afflittivo e sproporzionato rispetto all'offensività della condotta posta in essere dal soggetto agente avrebbe effetti deflagranti rispetto alla rieducazione del reo, poiché una pena disallineata rispetto alla condotta escluderebbe in radice un corretto percorso rieducativo e riabilitativo. Il disegno di legge governativo sembrerebbe sposare invece finalità o concezioni preventive della pena, a totale detrimento della funzione rieducatrice, dal momento che l'accento viene posto sulla necessità collettiva di sicurezza e stabilità.

Non ho interrotto prima che intervenisse il collega di Fratelli d'Italia. Tuttavia, signor Presidente, penso che sia importante, per l'Aula e per il Gruppo di appartenenza del sottosegretario Delmastro, ribadire un concetto. Noi, se il sottosegretario Delmastro si limita, signor Presidente, al parere conforme...

Il Gruppo Fratelli d'Italia ci deve dire se sta difendendo un uomo, un indagato o la loro idea di come si vive nelle istituzioni. Delmastro non solo è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio. Il sottosegretario Delmastro si è anche macchiato di un'offesa ad un'intera comunità politica. *(Commenti. che è cambiata la natura del suo Gruppo di appartenenza. Un tempo, di fronte a un reato così, sareste stati...

È evidente, signor Presidente, che le scuse non servono, se i comportamenti restano sempre gli stessi. Oggi voi avete dimostrato, tutti insieme, di non aver capito la gravità di quello che è accaduto. E non state offendendo, ancora una volta, il Gruppo Partito Democratico, ma un'intera comunità e la stessa Assemblea di Palazzo Madama. Signor Presidente, noi, ogni volta che il Sottosegretario prenderà la parola per esprimere un concetto, fino a quando non avrà affrontato il nodo, che è uno solo e che il senatore Bazoli ha ribadito, cioè fino a quando non avrà chiesto scusa alla comunità del Partito Democratico, usciremo dall'Aula e dalla Commissione. *(Applausi)*.

Signor Presidente, cari colleghi, trovo veramente inaccettabile che un Gruppo politico importante di quest'Aula, il cui rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche - a mio giudizio - fino ad oggi era al di sopra di ogni sospetto, possa permettersi in questa di voler imporre a un rappresentante del Governo di dire o non dire alcune cose. *(Applausi)*. Qualsiasi cosa essa sia, se il Gruppo PD si ritiene offeso dalle considerazioni del collega Delmastro Delle Vedove, ha tutti gli strumenti, dal giurì d'onore a una causa per diffamazione e a tutto ciò che in uno Stato di diritto è consentito, quanto previsto dalla Costituzione, a chi si ritiene leso in un diritto. Non ha invece alcun potere di imporre al Governo o a un suo rappresentante di dire o non dire, di fare o non fare alcune alcune considerazioni. *(Applausi)*. È un fatto gravissimo. Ritengo che sia un attentato alla Costituzione. E, se la vogliamo dire tutta, non spetta al Capogruppo del PD stabilire se Delmastro ha commesso o meno un reato. Tra l'altro, basta leggere la giurisprudenza relativa all'articolo 326 del codice penale per scoprire che non è punibile chi rivela un presunto segreto a chi ne ha diritto e non è discutibile che un parlamentare abbia diritto di accedere a quelle informazioni. Non è punibile il pubblico ufficiale che rivela un presunto segreto quando esso è di dominio pubblico e non è discutibile che c'erano giornali che già avevano pubblicato in quei momenti *(Applausi)* ciò che viene imputato a Delmastro di aver rivelato. Per cui, cari colleghi del PD, svolgete il ruolo il vostro ruolo con la capacità che tutti noi vi riconosciamo, con l'intelligenza che tutti noi auspichiamo, ma non ergetevi ad accusatori e giudici contemporaneamente. Non è un vostro compito. Per favore, lasciate intervenire il collega, come ho chiesto ai colleghi di Fratelli d'Italia di lasciare intervenire il presidente Boccia. BALBONI *(FdI)*. Concludo, Presidente. Io credo

pensavano, credevano e speravano di strumentalizzare Cospito per mettere in difficoltà il Governo Meloni, erano invece Cospito e, attraverso di lui, i mafiosi al 41-*bis* che strumentalizzavano il PD. Questa è la verità.

come dice giustamente il collega Borghi, ogni tanto parliamo anche nel merito. Vorrei soltanto annunciare che sugli emendamenti soppressivi il Gruppo Azione-Italia Viva voterà a favore per la soppressione per una questione di tipo tecnico. tecnico. Come abbiamo ampiamente discusso in Commissione, stiamo violando in modo patente il principio del *ne bis in idem*, e quindi, al di là della valutazione politica sull'opportunità o meno della norma, è ovviamente una norma che non sta in piedi e per questo voteremo l'emendamento soppressivo.

ha fatto una bellissima illustrazione delle ragioni di tutto l'impianto della normativa introdotta dalla legge n. 22 del 2022, cosiddetta legge Franceschini Orlando. Essa contiene non soltanto il danneggiamento, danneggiamento, ma anche norme che riguardano furto, autoriciclaggio e tutta una serie di condotte punite severamente, sulle cui ragioni difficilmente potrei spendere parole migliori di quelle che ha usato il collega Claudio Borghi nel ricordarci quanto dobbiamo difendere il nostro patrimonio culturale. Mi corre poi l'obbligo di leggere che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni culturali o paesaggistici propri o altri è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.500 va da sei mesi a tre anni più multa e la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose. Ohibò: è una norma che esiste già. Pertanto, a differenza di altre situazioni in cui ogni volta che c'è un problema c'è un riflesso automatico a creare una norma penale - questo sempre per il grande

quindi, è stato fatto un duplicato di norma con la sanzione amministrativa e questo è tutto il contrario di norme amministrative alternative al codice penale. è il motivo per cui noi presentiamo l'emendamento soppressivo 1.1. È fuori luogo discutere di quanto sia esecrabile imbrattare o deteriorare

anche con pene assolutamente elevate. Guardate che un altro mondo è possibile, cioè il legislatore può anche fare altro che non norme penali a raffica. Sono molti gli interventi per tutelare il patrimonio: si può intervenire socialmente, sono tante un po' di *relax* e fantasia, perché anche un po' di inventiva nel mondo che cambia non guasterebbe. Per questo chiediamo l'abrogazione dell'articolo

dato che siamo abituati ad avere nuovi reati ogni settimana, pensavo che fosse anche il turno dell'imbrattamento, e invece abbiamo trovato sanzioni amministrative. Poi naturalmente, aperto l'uovo di Pasqua, ci siamo accorti che c'era il verme dentro, nel senso che queste sanzioni amministrative vanno a a punire - come diceva la collega Rossomando - precisamente delle condotte che sono già previste e punite dal codice penale e vanno evidentemente a sovrapporsi con la sanzione penale. Senonché, in realtà devo riconoscere al collega Claudio di aver presentato un disegno di legge che invece aveva un senso, che è quello di andare a proteggere i beni strumentali alla fruizione dei beni culturali. Questo emendamento, quindi, serve a coprire quella lacuna che il disegno di legge del collega Borghi giustamente evidenziava, ma utilizzando non una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa, così dimostrando che possiamo reprimere fenomeni che creano allarme sociale senza ricorrere sempre alle manette e al diritto penale. Il tentativo che facciamo con questo emendamento, appunto, è di reprimere un fenomeno che va represso, perché è giusto che chi imbratta un bene strumentale, la fruizione del bene culturale, sia punito; ma per una volta possiamo dare la dimostrazione che utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione del legislatore e non la solita manetta, non la solita reclusione.

la sanzione viene applicata se è previsto che l'opera d'arte sia fruita dal pubblico. Per come era scritta la norma in precedenza, sostanzialmente, se il titolare di un'opera di cultura, che fosse però privata, non metteva a disposizione del pubblico il suo bene, incorreva nelle sanzioni previste. Avevamo statalizzato l'intero patrimonio culturale del Paese. Quindi, siamo intervenuti in Commissione, il Governo giustamente ha espresso parere favorevole e stiamo riallineando anche la norma del codice penale in modo tale che le due fattispecie siano identiche.

l'emendamento 1.0.103 mira a colmare un evidente *vulnus* del testo, laddove non prevede il consenso del condannato alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività.

Da ultimo, si ricorda che il consenso è elemento caratterizzante di tutte le ipotesi in cui sia prevista la sospensione condizionale, fatta eccezione per l'articolo in questione.

aggiungendo 10.000 euro di multa che, dal punto della politica criminale, non si capisce a cosa servano. Se la norma è afflittiva com'è, aggiungere 10.000 euro di multa sembra davvero un intervento singolare. Dato che la norma prevede già la reclusione fino a cinque anni, pensiamo che possa restare anche così e ci sembra già afflittiva abbastanza.

*In primis*, si sostituisce integralmente il testo dell'articolo 3 come approvato in Commissione; dopodiché, mediante la lettera *a)* si sopprime la condotta base di imbrattamento e la si trasferisce nel decreto legislativo relativo alle depenalizzazioni. similmente a quanto disposto per il danneggiamento che prevede la fattispecie base punita con sanzione pecuniaria civile e la condotta aggravata dalla violenza alla persona o minaccia ai sensi del codice penale, si prevede che nel codice penale sopravviva il comma relativo agli imbrattamenti dei beni immobili o sui mezzi di trasporto pubblici o privati, come modificata la lettera *b)* del presente emendamento. Da ultimo, con la lettera *c)* si elimina il riferimento alla procedibilità d'ufficio in quanto è stato eliminato il comma relativo alla condotta procedibile a querela.

come diceva Alberto Sordi, Roma non è una città come le altre: è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi. Ecco, io credo che in questa citazione, la capitale, Roma, possa essere tranquillamente considerata una sineddoche per tutta l'Italia ed è per questo motivo che per me intervenire oggi è motivo di orgoglio. Sono convinta, infatti, che il disegno di legge che stiamo discutendo sia di fondamentale importanza per il nostro Paese e per le future generazioni. Il patrimonio culturale ci è stato affidato dai nostri avi e in quest'ottica noi non ne siamo altro che custodi. Il nostro compito principale è garantirne l'integrità, in modo che possa goderne anche chi verrà dopo di noi. Il recente aumento di episodi di danneggiamento manifesta innegabilmente come ci sia bisogno di un'ulteriore stretta attraverso un deciso rafforzamento delle tutele che l'ordinamento presta ai beni culturali, che sono il vero patrimonio per cui l'Italia è riconosciuta nel mondo e che ne consente il posizionamento al vertice di tutte le classifiche, prima fra tutte quella dell'Unesco per ricchezza di patrimonio culturale e artistico. Sono anche contenta che l'esame di questa iniziativa legislativa prenda il via proprio da qui, dal nostro Senato, che solo pochi mesi fa è stato vittima a sua volta di un atto di becero vandalismo. Sì, è con cognizione di causa che lo definisco atto vandalico: quello che alcuni vorrebbero chiamare pacifica manifestazione di protesta non è altro che una forma di danneggiamento di un bene collettivo che si pone sullo stesso piano di coloro che deturpano i muri delle case, anzi peggio, perché il patrimonio culturale è un bene che coinvolge tutti noi, la nostra storia e la nostra tradizione. Ma non è solo per arginare questi cosiddetti fenomeni di attivismo del nuovo millennio che bisogna provvedere a inasprire il quadro sanzionatorio. Da decenni i nostri beni culturali sono vittima di atti di vandalismo che gridano vendetta al cielo e che sono motivati nei modi più disparati: dalla semplice bravata, alla protesta, alla semplice follia. Penso agli episodi avvenuti ai danni della Pietà o del David, entrambe opere di Michelangelo, ma più recentemente anche al lancio di colore sulla statua di Indro Montanelli, agli immancabili bagni nelle fontane capitoline, al deturpamento con incisione di una parete del Colosseo e ancora alla corsa con la Maserati giù dalla scalinata di Trinità dei Monti. Potrei citarne tantissimi, la lista purtroppo è tristemente lunga, ma credo che già questi esempi rappresentino sufficientemente bene il clima di emergenza che giustifica questo intervento che è volto sostanzialmente a proteggere il tessuto storico e sociale della nostra comunità di cui il patrimonio culturale rappresenta primaria manifestazione. Voglio quindi ringraziare il ministro Sangiuliano, anche se adesso non è qui presente, che prontamente e come non mai meritoriamente si è fatto portatore di queste istanze. Questi attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono da un lato danni economici ingentissimi alla collettività, che per il ripristino dei beni deve ricorrere all'ausilio di personale altamente specializzato specializzato e di macchinari costosissimi, ma al contempo attentano all'immagine del Paese, precludendo la fruibilità dei beni da parte della comunità nazionale e dei milioni di turisti che ogni anno decidono di passare del tempo nel nostro Paese per ammirarne la bellezza unica.

Se l'intervento legislativo del 2022, con cui sono state previste repressioni di tipo penalistico si è rivelato insufficiente, forse è anche perché tra misure alternative e sostitutive la reclusione non è più considerata un deterrente sufficientemente efficace. Confidiamo che il mutamento di prospettiva e l'introduzione di asprissime sanzioni pecuniarie possa contribuire alla tutela del nostro patrimonio culturale. Spetta a noi agire, a noi che in questo caso vogliamo rappresentare la stragrande maggioranza silenziosa di quegli italiani, di quelle persone per bene che amano il Paese e le sue bellezze e lo vogliono preservare dall'inciviltà di pochi. Proteggere il nostro patrimonio culturale significa proteggere la nostra storia, tutelare la nostra eredità per le future generazioni e in definitiva fare il nostro dovere. Per tutti questi motivi, con assoluta convinzione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole al disegno di legge in esame, con l'auspicio che possa essere un freno al ripetersi di incresciosi episodi che minano la nostra credibilità internazionale.

contro il corso di un'epoca che purtroppo ci sta facendo conoscere drammatiche emergenze. Se qualcuno dovesse analizzare la condizione sociale, ambientale e il contesto complessivo del nostro Paese attraverso gli atti che con tanta urgenza vi prodigate di portare in queste Aule, si farebbe l'idea di una comunità nazionale martoriata dal fenomeno dei *rave* illegali, sopraffatta dall'invasione di chi arriva nel nostro Paese fuggendo da guerre e disastri ambientali; si farebbe l'idea di un Paese oppresso da una schiera di imbrattatori seriali che mettono a repentaglio l'esistenza e la sicurezza del nostro immenso patrimonio artistico e culturale e in cui la GPA costituisce un comportamento di tale pericolosità e diffusione da giustificare la sua repressione tramite l'introduzione di un reato addirittura universale. Non c'è coincidenza, onorevoli colleghi della maggioranza, tra l'immagine del nostro Paese che costruite ad arte e il Paese reale, quello delle milioni di persone che ogni giorno hanno a che fare con problemi che continuate ad ignorare, nascondendoli sotto la cortina fumogena della paura e dei provvedimenti repressivi. Le vostre priorità politiche non coincidono affatto con quelle degli italiani, il distacco è clamoroso e questo provvedimento ne è l'ennesima dimostrazione. L'assenza di progettualità sui temi che stanno a cuore agli italiani, quelli che riguardano la loro qualità della vita, sembra coincidere con la vostra cultura profonda, che ha ancora il sapore delle vostre radici, autoritarie e fondate sul concetto che la repressione sia sempre e solo la soluzione dei problemi: la punizione come prima *ratio*. Non possiamo condividere questa impostazione, ovviamente. Il disegno di legge al nostro esame interviene aggravando un sistema sanzionatorio già esistente, nei confronti di gruppi specifici di oppositori, che esprimono dissenso attraverso atti non violenti. Questa è una scelta grave del vostro Governo, perché state di fatto facendo una legge *ad hoc* contro movimenti che esprimono opposizione, senza essere, di fatto, pericolosi. Si sta facendo una scelta di politica criminale, condannando questi attivisti che imbrattano con vernice lavabile opere del patrimonio culturale a pene sproporzionate ed esorbitanti, senza tener conto del complesso delle sanzioni già esistenti e contribuendo quindi a rendere farraginosa e disordinata la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, senza alcuna proporzione fra la gravità del comportamento e l'afflittività della sanzione. vi ricordo che quello di proporzionalità è un principio costituzionale e ha il valore di limite esterno al potere punitivo dello Stato. La politica rischia di guardare il dito e non la luna: il dito sono le azioni di protesta, la luna è il rischio di estinzione della specie. Di questo stiamo parlando, onorevoli colleghi, del rischio effettivo - se non cambiamo il corso delle politiche industriali e i nostri stili di vita - di vedere il genere umano sopraffatto dai cambiamenti del clima, che abbiamo prodotto noi umani e sui quali noi umani abbiamo il dovere di intervenire subito, prima che sia troppo tardi. I dettagli del disastro che ci attende non sono dati forniti da me, sono tutti nel *dossier* sui cambiamenti climatici pubblicato sul sito del Consiglio europeo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a leggerlo. Siamo sull'orlo del baratro, ma noi ci accaniamo contro chi butta vernice lavabile su un quadro o dentro una fontana. Dobbiamo avere paura di questo scenario, non della vernice sui muri. Certo, per la nostra cultura politica, le azioni di disobbedienza sono quelle di massa, quelle che portano alla partecipazione pubblica, ma quando vedo queste azioni più individuali, oltre a pensare ai beni presi di mira, non posso non pensare alle ragioni che portano questi ragazzi a compiere tali gesti, rischiando un processo. Mi interrogo sul perché e la risposta è che gli adulti hanno abdicato al proprio ruolo, non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto e quindi è naturale e sana la loro disperazione. Soltanto la disperazione può portare a un sacrificio così grande, tale da far rischiare un processo, il carcere e il futuro. Sbagliano le modalità? Certamente: i beni comuni non possono essere oggetto di deturpazione, ma ribadisco che il centro del tema non è e non può essere questo, se teniamo in considerazione il rischio concreto di cui stiamo parlando. Il rischio, onorevoli colleghi, è la fine del nostro pianeta. Per questo motivo, dichiaro il voto contrario al provvedimento sono passati per piazza Duomo, cioè quasi tutti, come succede a Milano, hanno trovato la statua equestre di Vittorio Emanuele II, quella grande, che sta proprio davanti al Duomo di Milano, coperta da una grande impalcatura. Perché c'è l'impalcatura intorno alla statua di Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo a Milano? Perché cinque persone lavoreranno, per un mese e mezzo, per per ripulire una statua che sarebbe stata sporcata con vernice lavabile. È talmente lavabile che ci vorranno 30.000 euro e cinque settimane di lavoro per rimetterla a posto. Ora, io ho il massimo rispetto per chi protesta e per chi lo fa per la conservazione dell'ambiente, ma deve essere molto chiaro che non è in questo modo che si manifesta per attirare l'attenzione nei confronti della preservazione del pianeta. È completamente sbagliato. Sarà che io sono romantico e penso a un tempo nel quale si protestava mettendo a rischio sé stessi, facendo lo sciopero della fame o sacrificando la propria persona, piuttosto che le opere d'arte, ma comunque questo è un modo di fare assolutamente non condivisibile. In questa sede, desidero esprimere la massima condivisione delle finalità, ma il massimo biasimo per gli strumenti che questi ragazzi utilizzano. Aggiungo il blocco del Grande raccordo anulare e tutto ciò che causa problemi non solo al nostro patrimonio artistico, ma anche alla vita delle persone che magari stanno andando a lavorare, in un ospedale o a fare cose che certamente non influiscono sulla salvaguardia del pianeta: di certo, impedire loro di farle non migliorerà la lotta per l'ambiente. Detto questo in premessa, per dire che, come Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, aderiamo allo spirito che guidava il Governo e la maggioranza in questo sforzo legislativo, questo disegno di legge è veramente un papocchio e una cosa inguardabile dal punto di vista giuridico e fa veramente impressione. Dovrò fare un grande sforzo per annunciare la nostra astensione, perché, nel leggere questo provvedimento, mi sento male. Si prende prende una norma che ne ricopia una del codice penale per introdurre una sanzione amministrativa, tra l'altro esosissima (perché parliamo di decine di migliaia di euro),

invece di rendere il processo penale più efficace e più celere, manda una bella cartella di Equitalia, bypassa tutte le garanzie che il processo penale prevede e che invece la cartella di Equitalia non prevede e così risolve la questione. Cari signori, caro sottosegretario Delmastro, caro ministro Nordio, non si fanno così le norme. Proprio non si fanno così. Questa è una norma che non si può votare, da questo punto di vista, così come non si può votare l'articolo 2, che - lo ripeto - lascia intonsa la norma com'era, aggiungendo 10.000 euro di multa. Mi chiedo, quando parliamo di cinque anni di reclusione, quale sia il *quid pluris* che ci porta a tale norma con questi 10.000 euro. Probabilmente il ministro Giorgetti è a corto di cassa e quindi, tra le multe e le cartelle di Equitalia, vuole migliorare il bilancio dello Stato; altrimenti, non si capisce che senso abbia, dal punto di vista legale e legislativo. Per quale motivo ci asterremo e non voteremo contro questa schifezza? schifezza? Sottosegretario Delmastro, lo dico a lei, che è qui: basta con un reato alla settimana, non ne possiamo più. Siamo partiti combattendo il panpenalismo, ma in Commissione giustizia abbiamo continuamente nuovi reati e nuove pene, ma non più soldi sulle carceri. Questo è il vostro paradosso: utilizzate di più le manette, ma non investite sulle case di reclusione e sulle case circondariali. Delle due l'una: o meno manette o più soldi sulle carceri, per aiutare anche la nostra Polizia penitenziaria. *(Applausi)*. Perché non voteremo contro e ci asterremo soltanto? Perché il collega Claudio Borghi, con il quale non sono mai d'accordo nella vita (ma si sa che anche gli orologi rotti fanno l'ora esatta due volte al giorno), questa volta ci ha visto giusto e si è accorto di un buco nella legge, quello della tutela dei beni strumentali alla fruizione dei beni culturali. Noi avremmo proposto una sanzione amministrativa, per evitare appunto il panpenalismo; però, dato che la norma effettivamente ha senso, perché va a coprire un buco, io direi che l'articolo 3 può essere votato (e infatti abbiamo votato favorevolmente). dalla risultante di due articoli che proprio non si possono guardare e di un articolo che invece di fatto va quantomeno a colmare una lacuna, se ne deduce che non ci può essere altro, da parte nostra, che un voto di astensione.

a vere e proprie aggressioni, motivate troppo spesso da furore ideologico. Mi vengono in mente i Buddha di Bamiyan, distrutti dai talebani. Mi vengono in mente la facciata e il proscenio del teatro di Palmira distrutti a mazzate da Daesh. Sono episodi che hanno colpito la nostra sensibilità e che, ahimè, Presidente, pur con connotazioni assolutamente diverse, abbiamo visto manifestarsi anche nel nostro Paese. Certo, non abbiamo avuto simili devastazioni, ma sicuramente vedere l'acqua della fontana di Trevi tinta di nero,

Da questo punto di vista, bisognava fare qualcosa e giustamente il Governo ha messo in cantiere il disegno di legge al nostro esame. Qualcuno ha detto che si tratta di danni lievi; no, non è vero, colleghi, perché in talune occasioni sono state usate sostanze lavabili, i danni permangono (sono stati anche citati poco fa in un intervento che mi ha preceduto) e i lavori per il loro ripristino sono di grande impegno economico. Bene quindi ha fatto il Governo a presentare questo disegno di legge, che intende perseguire con sanzioni, soprattutto di carattere pecuniario, in modo più impegnativo questi atti vandalici. L'idea è stata quella di introdurre sanzioni amministrative pesanti, aumentando le multe per chi deteriora beni culturali,

un comma che voglio annotare positivamente, perché si è andati a colpire la fattispecie del danneggiamento su su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, per evitare che rimanga privo di sanzione chi getta vernice o altro oggetto imbrattante su opere d'arte che pure sono protette per da un vetro o da altre strutture. Ad irrogare le sanzioni pecuniarie e amministrative ai trasgressori è chiamato il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione e, per evitare le censure relative alla violazione del principio generale del *ne bis in idem,* è stata introdotta una norma specifica, in base alla quale l'autorità giudiziaria - che probabilmente, per i tempi della giustizia, che notoriamente non sono brevissimi, interverrà successivamente a quella amministrativa - dovrà tener conto delle sanzioni pecuniarie e amministrative precedentemente irrogate. Ciò detto, Presidente, credo che la nuova normativa necessiterà di un monitoraggio, avendo evidentemente la finalità di scoraggiare questi atti di teppismo, di danneggiamento e di vandalismo; chiediamo quindi che poi ci sia un monitoraggio attento da parte del Ministero della giustizia - vedo qui presente il Sottosegretario - che dovrà verificare che le opere non vengano più colpite nel futuro, a seguito anche di queste sanzioni. Dall'altra parte, credo che dovremmo fare - e anche questo dibattito ritengo abbia una funzione positiva - un lavoro di mediazione e sensibilizzazione sul piano culturale nei confronti di chi adotta questo tipo di questo tipo di proteste in modo del tutto improprio, per far capire che non è questo il modo di far valere ragioni politiche che possono essere per certi versi apprezzabili, ma che non possono giustificare mai attentati di questo tipo. Ciò premesso, Presidente, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

questa nuova forma di protesta, nata a difesa dell'ambiente e ultimamente diffusa nelle principali città europee. Riguardo ai problemi del testo, veramente alzo le mani. Abbiamo fornito tutto il contributo possibile, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gli emendamenti presentati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle abbracciano l'intera struttura del disegno di legge, offrendo importanti spunti di riflessione dal punto di vista tecnico, al fine di attenuare lo scempio che avete avuto l'ardire di compiere. Il combinato disposto dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale (che ricordo essere attualmente vigente) e della disciplina punitiva operata per via amministrativa, che il Governo e la maggioranza intendono introdurre, renderebbe in maniera irragionevole enormemente afflittivo, forse sproporzionato e quindi incostituzionale il trattamento sanzionatorio che deriverebbe dal delitto di imbrattamento dei beni culturali. Sarà comunque il giudice delle leggi a valutare la corrispondenza del trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo* rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza sia nazionale sia eurounitaria, anche in ragione del rispetto del divieto *ne bis in idem.* Se ne dovesse derivare un giudizio contrario, non potrete dire che non ve l'avevamo detto. *(Applausi)*. La proporzionalità e l'adeguatezza della sanzione devono essere valutate anche in ragione dell'offensività della condotta posta in essere dal soggetto agente. Anche in questa sede ricordo che in giurisprudenza l'imbrattamento rappresenta un'alterazione temporanea e superficiale della *res*, il cui aspetto originale, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. Tali condotte, infatti, devono avere effetti rimovibili e quindi non devono incidere sulla funzionalità della cosa, in quanto, in caso contrario, sarà applicabile l'articolo 635 del codice penale, relativo al ben più grave reato di danneggiamento. Tanto doverosamente precisato, mi è dato rilevare come dopo nove mesi (quasi un anno di legislatura) ci sono questioni che ancora non mi sono chiare, come i pareri del Governo sugli emendamenti da noi redatti. redatti. La *ratio* con la quale il Dicastero si muove nell'espressione dei pareri mi è assolutamente oscura: come potete esprimere parere contrario a un emendamento che prevede la depenalizzazione della condotta base dell'imbrattamento, visto che il ben più grave delitto di danneggiamento semplice è stato depenalizzato nel 2016? Perché non prevedere l'esimente nei casi in cui l'imbrattamento possa essere eliminato all'istante e senza nessun problema da parte della persona che lo ha commesso? Perché non rivedere al ribasso l'impianto sanzionatorio, visto lo squilibrio che può ingenerare, se messo a paragone con le altre fattispecie, anche di più grave intensità delittuosa?

udite: prima si esprime parere contrario su un emendamento del MoVimento 5 Stelle, il relatore lo copia, *et voilà*, ecco il voto favorevole, fantastico! Cosa si farebbe pur di non dire quanto lavora bene il MoVimento 5 Stelle!

carbonica nell'atmosfera sembrano incontenibili, unitamente al riscaldamento della superficie terrestre; gli eventi climatici estremi sono purtroppo una logica conseguenza di questo inesorabile declino delle condizioni di vita del pianeta.

al fine di sviluppare una consapevolezza immediata della collettività relativamente al rischio che stiamo correndo. Ecco la consapevolezza che proprio gli autori di questi gesti cercano di farci acquisire. Nel corso della storia del nostro Paese sono stati diversi i movimenti di protesta che hanno caratterizzato momenti catartici, tutti accomunati da un'unica condizione, ossia che nel momento in cui sono stati posti in essere sono stati considerati come forme eversive di manifestazione del pensiero, ma a cui solo con una lettura a ritroso è stato dato il giusto peso. potrebbe questo fenomeno essere accomunato a quelli? Badate bene, non sto dicendo che il modo giusto per far intendere alla collettività il tema del surriscaldamento globale sia quello di imbrattare un quadro di Monet oppure di interrompere la gara dei 400 metri a ostacoli, rovinando per giunta anche la gara del corridore italiano Alessandro Sibilio, al quale va il nostro più sentito in bocca al lupo per una grandissima carriera, ma è il grido di una generazione che forse ha compreso ciò che noi ancora ci ostiniamo a non vedere. Il MoVimento 5 Stelle, anche in considerazione dell'obiettivo 2050, ha assolutamente a cuore i motivi della protesta e si batterà con tutte le forze a disposizione affinché la lotta al cambiamento climatico assurga a elemento caratterizzante di questa legislatura. Dalla nostra non abbiamo i numeri parlamentari per le battaglie che ci stiamo prefissando, ma ci batteremo anche per i movimenti che da fuori spingono per il medesimo obiettivo.

Noi ci faremo portavoce delle battaglie per la transizione ecologica portata avanti senza azioni a danno della collettività, anche perché il MoVimento 5 Stelle è nato proprio per battersi per difendere tali fondamentali valori. in conclusione, siamo contrari allo spirito di questa legge: aumentare scriteriatamente il trattamento sanzionatorio non avrà mai l'effetto di reprimere il compimento di determinate condotte, a maggior ragione se sono ancorate a ben saldi principi morali. azioni sbagliate, supportate da presupposti corretti. Per queste ragioni, dichiaro il voto fermamente contrario del MoVimento 5 Stelle.

la sospensione condizionale della pena o l'utilizzo della messa alla prova. Signori, dubito che vi siano persone che andranno in galera in applicazione di una delle norme penali previste oggi dal codice e bene ha pensato il ministro Sangiuliano di andare a intervenire invece in una maniera più diretta, che è difficilmente ovviabile, La sanzione amministrativa oggi quindi aggrava la posizione di coloro che danneggiano o imbrattano beni culturali e purtroppo sappiamo dalle notizie di giornale quanti sono i casi in

o danneggiamento viene commesso su teche, custodie o altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione dei beni culturali, questo comporti l'applicazione della pena della reclusione, nonché della multa. Dove questo disegno di legge è andato a intervenire

fra i vari, ricordo i vandali che hanno danneggiato la vetrata che protegge il Santissimo crocifisso della chiesa

agli Uffizi di Firenze, dei giovani si sono incollati al vetro; alla Cappella degli Scrovegni a Padova, due vandali si sono agganciati con le catene ai corrimano; ai Musei vaticani, alcuni ragazzi si sono legati alla base della statua del Laocoonte.

Dobbiamo rispondere con rigore e fermezza di fronte a queste manifestazioni. *(Applausi)*. Il disegno di legge in esame

le opere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico. Questo perché, signori? È ovvio che il bene culturale è un qualcosa che fa molto richiamo,

da parte dello Stato di fronte a eventi vandalici, che sono reati e magari vengono compiuti con la finalità di svolgere una manifestazione di dissenso per una questione climatica o quant'altro. Per noi restano solo reati. *(Applausi)*. La manifestazione dell'opinione può avvenire

tutti coloro che si stanno muovendo in queste direzioni, da chi sono finanziati? *(Applausi)*. La domanda è: chi pagherà le spese legali, chi pagherà il ripristino, chi pagherà le sanzioni?

Nell'ambito dell'associazione a delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, questi sono puniti a titolo di associazione a delinquere. Si ha un'associazione a delinquere quando ci si organizza per commettere un reato come quello del danneggiamento o deturpamento dei beni culturali. *Memento homo.* Grazie a voi tutti, colleghi, la Lega voterà convintamente a favore del provvedimento. Signor Presidente, per noi le rivendicazioni e le lotte che usino come strumento la deturpazione di un bene collettivo, a maggior ragione se di valore artistico, monumentale, culturale e ambientale, anche se ripristinabile a seguito di intervento, non rappresentano il metodo giusto per porre l'accento e la visibilità su quelle problematiche, anche di interesse generale. I ragazzi che hanno imbrattato i muri di Palazzo Vecchio, Palazzo Madama o la fontana della Barcaccia hanno compiuto per noi gesti sbagliati, violando norme già esistenti, e tra l'altro non raggiungono lo scopo che può essere essere alla base di certe rivendicazioni, ossia quello di creare consenso. Anzi, spesso producono una reazione opposta nell'opinione pubblica, che invece dovrebbe essere la prima degli alleati nelle battaglie di civiltà. Importa poco, insomma, se le vernici possono essere lavabili e se tutto può essere ripristinato, perché intanto lo si fa a spese della collettività. Credo che siano atti dovuti quelli compiuti dai sindaci delle città che hanno conosciuto queste cose.

assemblea - quelle delle centinaia di "angeli del fango" che nel 1966 salvarono i libri dall'alluvione di Firenze *(Applausi)* o di quelli che qualche settimana fa si sono rimboccati le maniche per aiutare a riparare i primi danni dell'alluvione, insieme alle donne e agli uomini delle città dell'Emilia Romagna. Detto questo, quei ragazzi hanno ragione nel merito delle questioni che, con metodo sbagliato, sollevano: chiedono di riappropriarsi del loro futuro, chiedono di farlo rivendicando un nuovo modello di sviluppo. Sono cose che si chiamano qualità ambientale, sostenibilità, giustizia sociale. Del resto, rendiamoci bene conto che il futuro è il loro, non il nostro. Sbagliano a imbrattare, ma ascoltiamoli. Rivendicano - com'è stato detto in questo dibattito - l'uscita dall'era dei combustibili fossili e più concretezza nell'affrontare la crisi climatica ed energetica; sanno che sta sfuggendo di mano anche al nostro Paese l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici. Che altro deve succedere oltre allo scioglimento dei ghiacciai, alle bombe d'acqua o al surriscaldamento di intere zone del pianeta? Quanti milioni sono i migranti climatici che fuggono e che fuggiranno ancora di più per insopportabili condizioni di vita, ma anche di lavoro in certe realtà vicino all'equatore? Che altro ci dicono i dati di ieri sulla mortalità degli anziani l'anno scorso in Europa e nel nostro Paese per il caldo? Mi stupisce - e lo dico con rammarico, senza particolare polemica - che i sostenitori della legge mettano l'accento sul contenuto specifico, ma ignorino completamente questo grido che con metodo sbagliato viene sostenuto. Nel merito, già i colleghi Alfredo Bazoli e Anna Rossomando hanno rappresentato bene la nostra contrarietà. Mi limito a riproporre in pochissimo tempo alcuni nostri rilievi molto seri. Per noi rappresenta un pasticcio sotto il profilo politico, giuridico e anche tecnico: questa legge, come quella sull'immaginaria emergenza *rave*, rientra in una strategia che è poi quella in senso lato del populismo penale. Quella sui *rave* in sede applicativa si è dimostrata una bolla di sapone; succederà anche in questa occasione. Anche i nostri Governi - pure questo è stato ricordato si sono occupati della tutela dei beni culturali, monumentali e ambientali. La legge denominata Franceschini-Orlando, per esempio, è stata una risposta seria perché organica, non una bandierina propagandistica, né un provvedimento *spot* adottato sull'onda di fatti di cronaca. Ugualmente organiche furono le norme approvate anni fa, sempre da parte di certe maggioranze da noi guidate e sostenute, sugli ecoreati, i reati contro l'ambiente, norme che anche stamattina, nel consueto rapporto annuale ecomafia di Legambiente, sono state ricordate ricordate e valutate come efficaci, serie e organiche. In Commissione abbiamo proposto emendamenti - non solo noi, ma anche altre forze di opposizione - per ridurre quello che per noi è un danno di questa legge, per modificarne l'impostazione, per migliorarlo, per attenuare le sanzioni e valorizzare anche una sorta di forma di giustizia riparativa. C'è stata sordità, sono stati respinti. Ciò la dice lunga sulla reale volontà che sta dietro questo atto. Per voi della maggioranza la cosa più importante sembra ossessivamente dare la percezione di una tolleranza zero, di un certo profilo giustizialista - sì, giustizialista - e ma inflessibile a giornate alterne, quando non interviene sui grandi interessi o su reati che sono davvero emergenze del Paese. Ne cito uno: il fenomeno della corruzione. *(Applausi)*. In sintesi, ho cercato di spiegare perché il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento.

Era il lontano 1922 e l'appena approvata legge sul paesaggio di Benedetto Croce introduceva una vera e propria svolta nella nostra legislazione ambientale. Secondo Croce l'ambiente e il paesaggio non erano altro che l'armoniosa convivenza e sovrapposizione tra elementi naturali, storici e artistici; detta più semplicemente, tra uomo e natura. Si tratta di principi tra essi complementari e non per forza antitetici, richiamati peraltro dall'articolo 9 della Costituzione, che oltre alle recenti integrazioni in tema di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, ricomprende la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. A dire il vero, Presidente, in tutto ciò qualcosa di antitetico e inconciliabile c'è eccome, ed è il cortocircuito generato da chi vandalizza il nostro patrimonio storico e artistico in nome dell'ambientalismo e la convinzione che la battaglia ecologista possa rimanere impunita nelle sue declinazioni prepotenti, irrispettose e dannose, una sorta di zona franca ideologica, che avanza sapendo di rischiare poco. poco. Non è così e non sarà più così: il provvedimento in esame oggi è una risposta forte e chiara che il Governo Meloni dà ai professionisti del degrado, con buona pace, sia chiaro, anche di quelle forze politiche che in cerca di facili consensi minimizzano o, peggio, strizzano l'occhio a tali dinamiche. Per quanto riguarda i contenuti, molto brevemente occorre sottolineare il duplice ambito di intervento: da un lato, vi è la necessità di rafforzare la tutela dei beni culturali o paesaggistici; dall'altro, quella di innalzare la soglia di attenzione a difesa dei beni pubblici e privati. In riferimento al primo punto, si introduce un secondo binario, che si affianca, pur senza intaccare il principio del *ne bis in idem*, a quanto già previsto dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale. Si tratta di sanzioni amministrative, che si aggiungono a quelle che verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile, ma con una differenza sostanziale: la tempestività. Sono infatti immediatamente erogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali, senza attendere quindi i tempi di avvio e di conclusione del procedimento.

ma è di salvaguardare gli interessi dello Stato e della collettività e di impedire che quel dissenso si traduca in prepotenza e in violenza a danno della comunità. Permettetemi di ricordare, in questo senso, quanto accaduto il 5 marzo scorso a Torino, prima capitale d'Italia, che si è risvegliata distrutta e devastata, profondamente ferita dal corteo anarchico che la sera e la notte precedente ha sfilato per le vie della città, a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime del 41-*bis*. Agenti contusi, cassonetti in fiamme, auto e vetrine distrutte, cartelli divelti, *dehors* devastati e interi palazzi imbrattati. Una città, tra lo sdegno generale, letteralmente messa a ferro e fuoco. Quanto andiamo ad approvare oggi lo dobbiamo a Torino, certo, ma lo dobbiamo a tutte quelle città che ospitano manifestazioni di qualsiasi tipo e natura, che si ritrovano a gestire, o meglio a subire passivamente, la guerriglia urbana causata dai soliti facinorosi. Auspico e ritengo che tali modifiche siano efficaci strumenti di deterrenza, nonché base di un rinnovato equilibrio tra interessi, di fatto non per forza divergenti. La protesta, intesa come sensibilizzazione, sollecitazione o critica costruttiva, va ricondotta all'interno di un patto di civiltà, di convivenza e di correttezza: è, in fondo, un elemento essenziale della democrazia e della cittadinanza attiva. Quando però essa travalica questi confini, sfociando in distruzione, guerriglia e prevaricazione violenta, lo Stato deve offrire una risposta ferma e decisa, ponendo fine all'epoca del permissivismo. Signor Presidente, il Governo Meloni proceda con coerenza, nel solco di quanto indicato all'interno del proprio programma elettorale, anche per ripagare la fiducia degli italiani, a più riprese confermata in questi mesi, e per rispondere alla crescente sensibilità in tema di legalità, sicurezza e ordine pubblico. Quanto ci apprestiamo a votare offre risposte concrete e puntuali in ma dirò di più: è la declinazione tangibile del concetto stesso di patria, a noi tanto caro. L'Italia, la nostra Patria, merita un sistema di regole che ne salvaguardi l'immenso patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, che ci rende unici in tutto il mondo. Gli italiani non chiedono solo rigore e norme più severe, a tutela del bene pubblico e privato. Gli italiani, eredi di chi ha reso la nostra Nazione ciò che è, pretendono che i nostri tesori, frutto di genio e instancabile lavoro, siano tutelati per le generazioni future e per questo meritano ascolto e rispetto. Tutti noi meritiamo un'Italia più giusta e responsabile e oggi compiamo insieme un altro piccolo passo in questa direzione. il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del provvedimento in esame.

in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale». *(Segue la votazione).*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

una grandinata devastante e imprevedibile, lo scorso giovedì 6 luglio, ha devastato un'ampia zona della Regione Piemonte, tra le province di Torino, Cuneo e Asti (la zona da cui provengo). grandine ha distrutto dal 70 fino al 100 per cento dei raccolti, senza contare i gravissimi danni ai fabbricati, alle aziende e agli automezzi; un evento davvero senza precedenti, con chicchi grandi quanto delle palline da tennis. Ho verificato io stesso i danni, nel corso di un lungo sopralluogo nelle zone colpite con gli assessori regionali, con il Governatore della Regione Piemonte, con il Presidente della Provincia, della Provincia, con i rappresentanti, i sindaci, gli amministratori, gli agricoltori e tutti coloro che hanno subito i danni. In particolare, le precipitazioni hanno insistito su Langhe-Roero, in provincia di Cuneo,

Si tratta, Presidente, di una grandinata senza precedenti, in un territorio che rappresenta un'assoluta eccellenza nel mondo per la produzione sia

visite agli ambienti e alle eccellenze della natura. Questo è un aspetto fondamentale e io sono qui oggi a segnalare a quest'Aula del Senato una situazione drammatica. Chiedo ai Ministri di competenza di attivare il Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi all'80 per cento - speriamo - dei danni subiti da coloro che non sono assicurati. Mi rivolgo anche alla Protezione civile, per un intervento sulle strutture fortemente danneggiate. Credo che sia il MASAF che il Dipartimento della protezione civile potranno dare manforte alla Regione Piemonte per avere a disposizione dei fondi. Spiace che si sia chiuso da poco il decreto alluvione, credo sia importante, perché c'erano delle misure che potevano contenere delle risorse immediate; è stata realizzata la cambiale agraria e sono state effettuate delle moratorie e delle sospensioni dei pagamenti

con il cuore pieno di tristezza, perché manca il raccolto, ma soprattutto perché in prospettiva, su certi tipi di colture come i vigneti, i noccioleti e i frutteti, i danni sono irreparabili per i prossimi due o tre anni. Esprimo pertanto da quest'Aula la solidarietà a tutto il territorio, ma soprattutto invoco la capacità di intervenire, di dare manforte e di aiutare economicamente queste zone devastate e questi imprenditori che hanno subito danni

Presidente, onorevoli colleghi, oggi prendo in esame la terza materia che costituisce la struttura portante di una società: quella dei trasporti e delle infrastrutture. ormai evidente che l'autonomia differenziata contribuirà ad aumentare la sperequazione fra Nord e Sud. La posizione geografica del Mezzogiorno assegna al nostro Paese una piattaforma logistica ideale nel Mediterraneo, sì da costituire una vera cerniera tra Europa, Africa e Asia. Non è un caso che nella classifica dei primi 20 scali europei per movimentazione *container* Gioia Tauro si posiziona all'ottavo posto, risultando lo scalo più importante del Paese, senza nemmeno essere servita da una infrastruttura ferroviaria adeguata. Purtroppo queste potenziali capacità di sviluppo vengono distrutte da una scarsa attenzione per migliorare i trasporti e le infrastrutture del Sud. Presidente, onorevoli colleghi, con l'autonomia differenziata si ridurrebbero ulteriormente gli investimenti nel Meridione. Addirittura nel Mezzogiorno negli ultimi anni si è disinvestito più di cinque volte rispetto al Centro-Nord. Secondo i dati forniti da Eurostat e rielaborati da Svimez, al 2016 nel Mezzogiorno per ogni 1.000 chilometri quadrati di superficie si registravano appena 18 chilometri di rete autostradale a fronte dei 30 del Nord e dei 20 del Centro. La stessa speculazione si registra anche per l'elettrificazione della rete ferroviaria; su 16.788 chilometri di rete l'elettrificazione delle infrastrutture meridionali sfiora il 50 per cento, mentre in altre parti d'Italia supera l'80 Tale sperequazione è ancora più evidente per l'Alta velocità. Questo ha portato il Sud a perdere l'occasione per assumere un ruolo predominante presso le rotte africane e asiatiche, impedendo all'intero sistema Paese e non solo al Sud di intercettare i flussi commerciali e turistici. Da questo Governo ci saremmo aspettati un impegno concreto per potenziare gli investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture così da connettere strade, porti scali, aerei e ferrovie, sfruttando anche a pieno le potenzialità della Via della seta, perché il commercio vuol dire, oltre che scambi di prodotti, soprattutto conoscenza, confronto ed inclusione, essere cioè messaggeri di pace. Qual è stata però la risposta di questo Governo? Il disegno di legge n. 615, la cosiddetta legge Calderoli, ciò che io chiamerei legge spacca Italia, che renderà l'Italia uno spezzatino di tanti staterelli. Noi del MoVimento 5 Stelle contrasteremo questo piano studiato a tavolino per dividere definitivamente l'Italia in due, un Nord opulento e un Sud colonia, assecondando il rigurgito secessionista e insensato della Lega di Gianfranco Miglio. Certamente noi non lo consentiremo. di contenuti tutelati dal diritto d'autore, approvato dalla Camera dei deputati; Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza; agricoltore custode dell'ambiente e del territorio; istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria; ripristino della festività nazionale del 4 novembre.

Grazie,